Ricordo che alle ore 12 il Ministro dell'interno renderà una informativa al Senato sui tragici fatti di Catania e sul fenomeno della violenza negli stadi. In quell'occasione il Presidente parlerà in ricordo dell'ispettore Filippo Raciti.

sono trascorsi appena tre mesi da quando questa stessa Assemblea è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti di costituzionalità del decreto n. 261, il quale l'attuale Governo affrontava la spinosa questione della sospensione delle procedure di sfratto per particolari categorie socialmente deboli. Come noto, in quella occasione il Senato, con 151 voti a favore e 147 contrari, decretò la fine di un provvedimento iniquo ed incostituzionale sotto più profili. Ed infatti, nel testo del decreto erano nascoste numerose disposizioni insidiose che creavano disparità di trattamento inaccettabili e configuravano, per alcune fattispecie, un vero e proprio esproprio del diritto di proprietà, oltretutto privo del relativo indennizzo costituzionalmente prescritto. Così che, seppure nelle dichiarazioni dei proponenti il provvedimento era stato varato per far fronte all'impossibilità delle forze dell'ordine (già impegnate in numerosi compiti prioritari di impegni quali esiti dell'indulto e sorveglianza di obiettivi sensibili) di occuparsi anche delle esecuzioni dei decreti di sfratto, nella realtà, si era rivelato lo strumento con il quale venivano accolte le ragioni della componente di estrema sinistra del Governo, le cui rivendicazioni, come noto, tendono a colpire innanzitutto la proprietà immobiliare che, secondo qualche esponente della sinistra stessa, dovrebbe addirittura essere requisita. Fra le varie disposizioni del vecchio decreto-legge, chiaramente anticostituzionali, come denunciato dai colleghi Pastore e Ferrara nella pregiudiziale, era particolarmente rilevante quella che *ope legis* riconosceva il diritto di rinnovo per nove anni del contratto scaduto in caso di unità immobiliari oggetto di cartolarizzazione, con devastanti conseguenze anche sulla possibilità di attirare investimenti italiani ed esteri nel settore immobiliare. Benché l'attuale disegno di legge abbia quindi dovuto stralciare questa assurdità, a me pare tuttavia doveroso rimarcare il tentativo iniziale perché, una volta di più, sia chiaro come nel DNA di questa sinistra sia preminente l'istinto preventivo specialmente della piccola imprenditoria privata, in contrasto con le dichiarazioni mediatiche di liberalizzazioni e quant'altro. Riconosco ovviamente che il presente disegno di legge tenta di risolvere il problema reale del disagio abitativo di categorie socialmente deboli, ma ciò non può essere fatto introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di locatori, stanziando poche risorse (63 milioni di euro), scaricando il problema sui Comuni e prevedendo scarsissime agevolazioni fiscali verso proprietari che subiscono o aderiscono alla proroga. Rimangono, inoltre, nel disegno di legge talune criticabili disposizioni, quali l'allargamento del beneficio ad attività teatrali,

familiare interessato abbia la presenza di un ultrasessantacinquenne e/o un figlio fiscalmente a carico, anche ventottenne; il che vuol dire praticamente nessuno escluso!). Ciò detto, è prevedibile che prossimamente nascerà la necessità di altra proroga, in quanto le misure adottate non offrono capacità di suscitare anche iniziative imprenditoriali private in questo campo, seppur di piccola entità, ma molto diffuse. Infatti, prima di iniziare le procedure localmente da parte dei Comuni, sono previste una pletora di tavoli di cosiddetta concertazione, a livello parlamentare, ministeriale, regionale, sindacale, ANCI, eccetera, sicché i tempi effettivamente necessari saranno infruttuosamente superati. Concludendo, a parte la proroga degli sfratti condivisibile e necessaria, questo disegno di legge in prospettiva non risolverà il problema del disagio abitativo delle categorie deboli, ma riuscirà benissimo a far progredire il processo di penalizzazione dei diritti, specie dei piccoli proprietari, umiliandone l'iniziativa, e proseguendo nel percorso messo in campo, come a tutti noto, nella contestatissima finanziaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'ordine del giorno da me presentato e che mi appresto ad illustrare prende le mosse da una particolare condizione di disagio abitativo che, pur non rientrando nelle fattispecie previste dal provvedimento all'esame dell'Aula, è comunque meritevole di attenzione e di specifico interesse da parte del Governo. Trattasi della situazione che vede coinvolte, soltanto nella città di Livorno, circa 680 famiglie, costituitesi ormai da più di un decennio in apposito comitato, detto degli esclusi, le quali si trovano da anni nella paradossale condizione di non vedere riconosciuto il proprio diritto all'acquisto dell'immobile, né il proprio *status* di conduttori affìttuari.

1993, 19 alloggi con più di 50 anni dalla loro realizzazione che, solo per questo fatto e non per un particolare pregio architettonico degli edifici, sono risultati inalienabili in quanto soggetti alla tutela dei beni culturali, ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Tra l'altro, gli immobili in questione sono per lo più in condizione di accentuata obsolescenza e bisognosi di profonde ristrutturazioni, cosa questa che rende le condizioni di vita degli inquilini in un evidente stato di disagio, precludendo loro la possibilità di interventi diretti tesi alla ristrutturazione, in quanto non proprietari; ma al contempo disincentivando la proprietà (ieri la Regione e per essa l'ATER, oggi il Comune) ad effettuare interventi su immobili per cui resta valido il programma di alienazione. Con questo ordine del giorno si intende pertanto porre, una volta di più, all'attenzione del Governo la questione in oggetto, chiedendo al riguardo l'opportunità di assumere le adeguate iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui attuale definizione, come ho cercato succintamente di illustrare, ha prodotto in talune circostanze contenziosi e ingiustizie. Il presente ordine del giorno si giustifica anche in ragione del carattere di organicità che il provvedimento in approvazione riveste, costituendo, rispetto al passato, un segnale di forte discontinuità, tanto da prevedere specifiche azioni tese ad avviare il problema abitativo a soluzione, sia con un piano straordinario pluriennale da parte dei Comuni, sia con un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica da parte dello Stato.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, noi sosterremo e sosteniamo senza riserve, ma con grande preoccupazione sullo stato delle politiche abitative, la veloce approvazione del disegno di legge oggi alla nostra attenzione, che consente il blocco degli sfratti per le famiglie con un reddito inferiore a 27.000 euro e carichi familiari e sociali che determinano gravi difficoltà. La decadenza del precedente decreto, nel passato autunno, ha già posto in drammatica discussione la serenità di migliaia di famiglie. La grande preoccupazione è data dall'oggettiva constatazione, che oggi entra nella norma, che con 1.200 euro mensili è diventato impossibile prendere casa in affitto. Se questa legge è quindi un atto dovuto, che tampona, con ritardo, una grande emergenza sociale, vogliamo cogliere in questo provvedimento un primo anticipo di una politica complessiva per la casa, politica quanto mai urgente, visto l'evidente rischio che la situazione si incancrenisca drammaticamente. Già la scelta dell'obbligo per i Comuni di prendere atto con serietà del drammatico problema attraverso specifici piani triennali è un primo passo importante. L'impegno del Governo a superare la pratica della proroga periodica, come richiesto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2004, passa attraverso la piena consapevolezza che il tema di cui dibattiamo necessita di una profonda riflessione sul rapporto tra pubblico e privato: la mano invisibile del mercato, sul terreno immobiliare, ha drammaticamente fallito, e oggi non solo ci troviamo a tamponare situazioni di emergenza, ma anche a interrogarci sulla sostenibilità dei costi della casa per fasce ben più larghe di quelle tradizionalmente ritenute deboli. Questo provvedimento è necessario, ma non esaurisce il tema complesso che abbiamo di fronte e rischia di essere inutile se non si assumono ulteriori impegni: occorre invertire la tendenza a non programmare, a non intervenire sul sistema degli affitti, a non agire per l'edilizia pubblica. Se nel nostro Paese il 78 per cento delle famiglie ha una casa in proprietà, si calcola tuttavia che 4 milioni di italiani abitano in affitto e ben 600.000 sono le domande per ottenere una casa popolare. Sempre più difficile risulta trovare casa in affitto per il rincaro dei prezzi non più sopportabile, in particolare dai giovani e dai lavoratori precari, che spesso non possono neppure accedere ai mutui per l'acquisto. Se, come ci dice l'ISTAT, il 70 per cento dei giovani tra i 20 e i 34 anni vive ancora sotto il tetto dei genitori, non è certo per un eccessivo affetto familiare, ma per l'impossibilità materiale di costruirsi un percorso autonomo di vita. E ancora, come non ricordare la denuncia dello stesso Ministro dell'interno relativamente alla pratica vergognosa dell'affitto in nero di alloggi, soprattutto a lavoratori immigrati, regolari e clandestini, ammassati in 10 per stanza? Siamo di fronte dunque ad una emergenza casa, ed è bene averne piena consapevolezza. Una emergenza che l'irresponsabilità di chi ha scelto di giocare la politica sulla pelle dei cittadini ha reso, con la decadenza del precedente decreto, ancora più grave. E deve essere chiaro come le cartolarizzazioni degli immobili degli enti siano state un duro colpo al diritto alla casa, in solo favore della rendita. Cogliamo con soddisfazione una proroga ulteriore e rafforzata per i grandi patrimoni immobiliari: in questo modo riaffermiamo come la casa sia prima un diritto e solo dopo un mercato. Per questo occorre quel cambiamento nella politica della casa che ha annunciato il Governo. La proroga degli sfratti è accompagnata da un tavolo di lavoro e, soprattutto, da un impegno serio per interventi sugli affitti e per incrementare l'offerta adeguandola alle nuove tipologie, alla domanda reale. Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, siamo certi che il Governo continuerà la concertazione che è stata avviata. Occorre concertare un piano nazionale e porre a disposizione le necessarie risorse; occorrono investimenti per l'edilizia popolare nelle forme che si rendono più efficaci. In questa sede, la più autorevole, come è il Parlamento, affermiamo il nostro appello affinché questa sia considerata una priorità sia dal Governo che dalla maggioranza. Per quanto riguarda il rapporto con le autonomie locali, indispensabile in questa materia, non si tratta solo di concertare gli interventi e di ottimizzare le risorse, ma occorre rendere nuovamente centrale l'urbanistica, come capacità di governare il territorio per il bene comune. Ogni qual volta si è liberalizzato l'uso del suolo si sono arrecati danni ambientali talvolta irreparabili e si è sacrificata sull'altare del profitto dei soliti noti l'edilizia popolare. Già oggi cogliamo segnali positivi, anche per gli effetti che la politica immobiliare ha per il tessuto sociale: si pensi alla prima riflessione sul ruolo della cultura nelle città con l'intervento che oggi approviamo sui teatri. Il Governo, in coerenza con il programma dell'Unione, sa bene non solo che si tratta di superare l'incuria degli anni più recenti, ma anche che una politica per la casa non può essere incardinata su vecchi modelli: oltre alle esigenze della cosiddetta famiglia tradizionale, si presentano le richieste, le esigenze di parti della popolazione che trovano grandi difficoltà a veder garantito il diritto alla casa ed in particolare i giovani, le coppie di fatto, i *single*. Occorre dunque calibrare per aree geografiche, struttura sociale, tipologie abitative; una nuova politica della casa che abbia i connotati di un grande investimento sul futuro del Paese e sui giovani in particolare. In conclusione, ribadendo la nostra posizione favorevole su questo intervento, affermiamo l'impegno sui seguenti chiari obiettivi: intervenire sulla legge che regola gli affitti in modo da far emergere il sommerso, anche agendo sulla leva fiscale; ridare slancio all'edilizia residenziale pubblica contrastando, con misure adeguate, la liberalizzazione dell'uso del suolo. Superare, dunque, la ripetitività delle proroghe degli sfratti, affrontare in modo organico l'emergenza sociale della casa e dare corso agli impegni chiari e convincenti

Presidente, comincerei in modo molto banale e semplice: è facile dire - ed è giusto dire - che ognuno e ciascuno ha bisogno di una casa. Una casa che è un luogo fisico, ma è anche un luogo mentale che ci che ci parla di appartenenza, sicurezza, benessere, relazioni e, infine, della propria identità. Nel nostro Paese è mancata da almeno due decenni a questa parte una seria ed efficace politica sociale della casa, capace di dare soddisfazione ad un bisogno, che è un diritto, che la precarietà del lavoro, le nuove povertà, la vulnerabilità sociale, il cinismo legislativo hanno reso impellente e che segnano drammaticamente le nostre città, piene degli spazi lasciati vuoti dalla produzione industriale, che si sono riconvertiti a produzione del disagio, di emarginazione e di degrado. Chi stava al Governo nella passata legislatura aveva fin dalla sua costituzione nominato il tema ma, ciò nonostante, abbiamo visto alienazione del patrimonio pubblico, cartolarizzazioni e uso dissennato del territorio.

Quelle immagini sono appunto un simbolo e ci paiono legate, anche emotivamente, all'avvento del nuovo corso politico, capace - vogliamo sperare e, per questo, lavorare - di fronteggiare tra l'altro la speculazione immobiliare e l'uso rapace del territorio, capace di far risuonare nelle istituzioni, anche le più alte, che a volte sono anche le più distanti, la voce dei bisogni delle persone, dei cittadini e delle cittadine di quelle fasce sociali più deboli sul mercato, avviando un percorso di presa in carico delle problematiche più urgenti e più dimenticate, come quelle della casa, della qualità del vivere e dell'abitare, che hanno a che fare anche con la qualità della vivibilità urbana. al problema della casa in Piemonte, in particolare a Torino, i dati sono molto forti e interessanti: sono state 8.500 le domande per l'assegnazione di una casa popolare presentate lo scorso anno,

è un *trend* (8.000 domande) in crescita, un fenomeno in fase di espansione. I dati più significativi sono la tenuta delle domande dei richiedenti nati in Italia, una flessione di quelle presentate da persone originarie del Maghreb e da famiglie provenienti dall'area dei Balcani, mentre in aumento sono quelle dell'Est europeo. È poi in aumento la gravità del disagio abitativo. I richiedenti hanno un punteggio più alto, quindi si è verificato un peggioramento delle condizioni denunciate. Il 40 per cento del disagio abitativo grave è legato alle condizioni della casa: sei su dieci domande rivelano sovraffollamento. Nel 40 per cento dei casi c'è una situazione reddituale estremamente grave, mentre il 79,8 per cento presenta una situazione medio grave.

I richiedenti con meno di 40 anni di età rappresentano il 42 per cento sul totale dei partecipanti, mentre l'incremento delle domande di giovani con meno di 30 anni è pari all'80 Sono dati molto forti e significativi. Riteniamo che con il disegno di legge n. 1231 si stia avviando un processo positivo per affrontare la complessa tematica del disagio abitativo. Infatti, nel provvedimento si prevede non solo la proroga degli sfratti per le categorie esposte ad una maggiore fragilità sociale, ma pure l'avvio di un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata ed agevolata. La questione è complessa e necessita di risposte differenziate: dalla messa a disposizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata allo sviluppo di interventi per favorire l'offerta di alloggi a canone sociale e al sostegno ai cittadini e alle cittadine con l'utilizzo del Fondo sociale per la casa. E' auspicabile e necessario che le politiche per la casa si integrino con le politiche urbanistiche volte al recupero dei centri storici e delle periferie. In Piemonte, a Torino in particolare, il perdurare della crisi industriale e manifatturiera, le trasformazioni del mercato del lavoro e delle diverse forme di organizzazione della produzione e quindi del sociale, i mutamenti demografici hanno aperto, accanto al problema delle persone in situazione di povertà, un nuovo fenomeno sociale: quello della vulnerabilità sociale. Accanto a chi vive in miseria, perché privo degli elementi essenziali che assicurino condizioni di vita sufficienti, vi sono cioè i cosiddetti nuovi poveri, quei soggetti che, in conseguenza delle politiche di mercato, cadono nella rete della povertà, che diviene stabile per carenza di strumenti. Per queste persone e per queste situazioni la mancanza di una casa diventa un elemento di caduta sociale drammatico. La Regione Piemonte ha tentato di fronteggiare questa situazione di grande emergenza sociale predisponendo un programma pluriennale per l'edilizia popolare 2006-2012, per il quale i finanziamenti coprono solo il biennio 2007-2008, anche a causa delle politiche iperliberiste del precedente Governo, che aveva ridotto notevolmente i finanziamenti per l'edilizia pubblica fino ad arrivare a prevedere zero finanziamenti per il settore per l'anno 2004. Il provvedimento in discussione oggi tenta di superare la mera proroga degli sfratti fine a se stessa e prevede che tale sospensione sia finalizzata all'effettivo avvio di programmi per la soluzione del problema abitativo delle categorie interessate. Il Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sostiene questo provvedimento, ma non vanno sottaciute le perplessità sull'insieme delle politiche per la casa. Ribadiamo che alle politiche abitative va assegnata una priorità nazionale. Il *trend* in atto e i presumibili sviluppi futuri stanno progressivamente facendo emergere nuovi bisogni ed aree di disagio abitativo, concentrati nei segmenti sociali ben definiti rappresentati, come dicevo prima, da lavoratori atipici, famiglie monoreddito, anziani, lavoratori in mobilità, studenti e migranti. Bisogna rendere, per questo, più efficaci i sostegni finanziari alla domanda, ristabilendo una fonte di finanziamento certa, stabile e adeguata al fondo di sostegno per le famiglie in affitto con difficoltà. Si tratta di una questione che le ultime leggi finanziarie hanno pesantemente penalizzato e che nemmeno la legge finanziaria 2007 ha affrontato in maniera adeguata, perlomeno nello stanziamento di risorse. Per questo diamo molta importanza alla convocazione del tavolo di concertazione tra Governo, Regioni e Comuni per l'individuazione di un piano pluriennale nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, anche mediante l'acquisizione, ristrutturazione o manutenzione di edifici esistenti, finalizzato all'aumento di alloggi in locazione a canone sociale da canone concordato. Anche in questo modo si combatte la crescita dei prezzi degli affitti. Infine, crediamo che il mercato degli affitti privati possa essere moderato anche attraverso lo strumento degli incentivi fiscali, incrementando la detassazione degli affitti a canone concordato. Sulla casa siamo ad un punto di svolta: il tavolo nazionale sulla concertazione, di cui dicevamo prima, può diventare una specie di «stati generali» per il diritto alla casa, con un ruolo attivo degli enti locali, delle Regioni, dei sindacati e del movimento per la casa.

nella materia del contratto di locazione e del blocco delle esecuzioni per sfratto.

fino al recente passato, è stata smantellata per dare finalmente luogo ad un mercato delle locazioni sufficientemente libero, quindi rimesso alla determinazione dei canoni sulla base della domanda e dell'offerta, senza

segnato la via maestra per il legislatore la giurisprudenza della Corte costituzionale che, prima con enunciazioni di principio e poi anche con dichiarazioni di illegittimità costituzionale di decreti-legge e di provvedimenti

la normazione in materia di sospensione dell'esecuzione deve riguardare un periodo transitorio ed essenzialmente non illimitato; bisogna poi tenere in carico alcune valutazioni comparative tra la situazione di disagio del conduttore ed eventuali situazioni di disagio dello stesso locatore; indicava come punto di riferimento per una possibile soluzione del problema del disagio abitativo il ricorso a strumenti che ponessero in carico il problema all'intera collettività non soltanto ad alcuni singoli soggetti che per ventura si fossero trovati a dovere alleviare con un sacrificio economico personale le situazioni di disagio in cui si trovavano i conduttori degli immobili di proprietà di questi soggetti.

e individuando categorie di disagio ben definite per qualificare e per dotare questi soggetti di particolari garanzie. Ricordo anche brevemente che questo disegno di legge fa seguito a un decreto-legge presentato dal Governo che ha subito in quest'Aula un fermo sulla base di presupposti di costituzionalità. Per questo motivo è importante verificare se anche il disegno di legge in esame ha le stesse caratteristiche in negativo. Quali furono all'epoca le motivazioni portate in questa sede sulle quali si basò il voto favorevole alle pregiudiziali da parte dell'Aula? la prima, il decreto‑legge ampliava notevolmente la platea del territorio al quale applicare questa normativa speciale,

in maniera formale indicare dei meccanismi selettivi, ma in maniera sostanziale non indicare alcuna selezione. Infatti, quando il decreto‑legge di allora decaduto parlava dei Comuni capoluogo di Provincia e di Comuni limitrofi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in realtà indicava una mappatura territoriale che comprendeva la maggior parte del territorio italiano. Non solo, ma alle nostre richieste di

dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa. Ricordo che tale elenco viene aggiornato e quindi fotografa la realtà viva del nostro Paese e non si ferma ad indicazioni

per il quale, ripeto, non trovo giustificazioni, vista anche la varietà del nostro quadro delle Province italiane (si va da Province con milioni di abitanti a Province che non arrivano forse nemmeno a 150.000 abitanti)

solo a soggetti privati che possono trarre da un certo numero di immobili un'aspettativa nella gestione del loro conto economico e dei loro equilibri finanziari

che, dalla redditività degli immobili e dalla possibilità di ottenere un rilascio certo e comunque non discriminatorio rispetto a a quello stabilito per tutti gli altri proprietari, traggono ragione di un equilibrio economico che è interesse di tutti conservare.

e rendere autosufficienti nella gestione delle loro importanti funzioni di livello pubblico anche attraverso una corretta redditività del loro patrimonio. Questa norma, una norma chiaramente demagogica, è rimasta anche nel disegno di legge al nostro esame e non può che gettare incertezza nel campo immobiliare, perché è evidente che chi gestisce o

tenendo conto che per i piccoli proprietari in situazioni di disagio ci si trova di fronte alla possibilità - proprio sulla base di quell'esigenza di comparazione tra necessità del conduttore e del locatore - data ai privati di - data ai privati di poter addirittura ottenere il rilascio in caso di situazioni analoghe a quelle del conduttore, mentre è chiaro che questa possibilità non si proporrà mai per i grandi proprietari. Mi sembra appunto una

o ritenute esistenti da una parte politica diverse condizioni economiche di un soggetto rispetto a un altro, pur essendo in un sistema di mercato libero.

Oltre a quanto ricordato finora, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula e del Ministro un paio di questioni sostanzialmente nuove rispetto a quelle che ho indicato e che riguardano anche profili inerenti alla lettura della legge, e quindi alla sua legittimità, perché potrebbero portare tale lettura a debordare i limiti posti dalla Corte costituzionale. Mi riferisco all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1.

nella parte iniziale dello stesso comma: da ciò derivava che la presenza nel proprio nucleo familiare di figli fiscalmente a carico costituiva una di quelle condizioni di disagio abitativo che poteva dar luogo, unitamente al reddito inferiore a una certa soglia e all'impossidenza di altra casa adeguata, all'applicazione di questo blocco. La Camera dei deputati ha inventato questa formula,

perché si abbia il blocco degli sfratti: basterebbe dunque la presenza di figli a carico, naturalmente nei Comuni previsti nella prima parte del primo comma, perché si applichi il blocco

giacché la norma sul prolungamento della durata dei contratti che hanno per oggetto questo tipo di immobili si applica non solo alle proroghe dei contratti in essere, ma anche

sulla legittimità costituzionale dell'articolo 7, al di là del merito e quindi dell'ampliamento della tipologia contrattuale prevista per gli alberghi agli immobili agli immobili destinati ad attività teatrali. Desidero far presente ai colleghi che non abbiamo voluto tradurre queste obiezioni in una pregiudiziale di costituzionalità

della prima abitazione, cioè della casa in cui vivono. Ciò è dovuto anche all'aspettativa di un mercato libero, che ha permesso a molti che pensavano di poter godere di vincoli ultradecennali della legislazione precedente di capire che la casa è un bene che deve essere acquistato sul mercato.

ma si ispira assolutamente agli stessi scopi, cioè contenere il disagio abitativo, l'emergenza del problema casa (ne ha parlato molto bene prima la collega senatrice Alfonzi, quindi non ci torno su), un'emergenza drammatica nella nostra società.

la sospensione finalizzata alla conclusione di iniziative che possono in seguito dare luogo a dismissioni per quegli alloggi - qui è la particolarità dell'ordine del giorno «siti all'interno di strutture non operative (con ingressi separati) gestiti dal Ministero dell'interno». L'oggetto di cui si tratta sono alloggi del demanio che il Ministero dell'interno ha concesso in uso a titolo oneroso ai suoi dipendenti

regolarmente inquilini fino al 1999, quando poi è stata sospesa bruscamente la riscossione dei canoni, a cui sono seguite le istanze di recupero forzoso (gli sfratti). Noi chiediamo la sospensione degli sfratti per questi soggetti e, in analogia a una risoluzione che è stata adottata in Commissione difesa alla Camera il 4 ottobre 2006, quindi recentemente, che la prevedeva per i soggetti dipendenti dell'Amministrazione della difesa, crediamo che questa tutela vada estesa anche ai soggetti dell'ordine del giorno in questione, per una ragione anche di di attualità: abbiamo manifestato in questi giorni grandissima solidarietà alle forze di pubblica sicurezza per i tragici fatti di Catania alla famiglia di Filippo Raciti, e quando si tratta delle cause di morte per servizio facciamo spesso molta, troppa demagogia, ma facciamo molta fatica a riconoscere i diritti sociali

ma che debbano sapere che noi li consideriamo parte del mondo del lavoro, con problemi e disagi simili a quelli degli altri lavoratori e che per questo intendiamo tutelarli.

il disegno di legge n. 1231, inerente «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», è di grande importanza politica e rappresenta uno dei principali provvedimenti, a mio avviso, che evidenziano

a prorogare gli sfratti, pur sulla base di precisi criteri sia territoriali che di condizioni socio-economiche delle famiglie, ma risponde a una forte attesa sociale legata a precise emergenze, su cui tornerò brevemente; soprattutto - ecco la novità apre una stagione nuova di politica abitativa riferita, in particolare, alla locazione dei ceti più deboli, come ha opportunamente evidenziato nella sua relazione il senatore Confalonieri. Non si tratta di una proroga di otto mesi fine a se stessa; nel disegno di legge, infatti,

In Italia, oltre 600.000 famiglie sono nelle graduatorie per l'acceso alle case popolari. Ciò avviene perché si costruiscono sempre meno alloggi popolari:

famiglie possiede la propria casa, ma non può essere l'unica soluzione, perché è la causa, tra l'altro, di enormi indebitamenti per l'acquisto della prima casa. Insomma,

È una politica non solo antipopolare, ma sbagliata, direi poco moderna e non europea, se è vero che oggi gli alloggi sociali in Italia rappresentano solo il 4 per cento (lo ricordava sempre il senatore Confalonieri) del patrimonio edilizio, mentre in Europa la media è del 16

un piano nazionale per l'edilizia pubblica residenziale: il comma 1154 della finanziaria individua risorse pari a 60 milioni per il prossimo biennio, ed è solo un avvio. Ringrazio molto il ministro Ferrero che, sin dalla prima versione del decreto-legge, aveva posto

Va quindi riproposto il tema del finanziamento pubblico per l'edilizia sociale e del diritto alla casa come uno dei principali diritti di cittadinanza. Su questo aspetto ci uniamo ai movimenti, ai comitati degli inquilini e ai sindacati dei lavoratori. C'è un nesso molto positivo fra la norma introdotta in finanziaria,

i Comuni e le Regioni devono definire i piani straordinari. So che ci si sta muovendo in tale direzione anche nella città da cui provengo, Napoli, certamente una delle capitali del disagio abitativo: nel quadro di quasi 10.000 sfratti

Proprio noi, che abbiamo espresso gravi preoccupazioni per il ritardo di questo provvedimento e per la drammaticità della condizione dell'emergenza abitativa, ribadiamo che non bastano solo provvedimenti emergenziali. Siamo molto contenti del provvedimento in esame proprio perché si inizia finalmente a riparlare di politiche strutturali in grado di dare certezze sia agli inquilini che ai proprietari.

È chiaro che, a fronte di questa ritmicità, è difficile continuare a parlare di emergenza. Nella passata legislatura abbiamo manifestato scarso entusiasmo per i decreti che puntualmente ogni anno ci venivano proposti, con motivazioni diverse, per prorogare le condizioni per il rilascio al proprietario di un alloggio in affitto a favore di particolari categorie sociali. Questo atteggiamento non era certamente dettato da scarsa consapevolezza sulle ragioni solidaristiche del provvedimento, quanto dal rifiuto di accettare l'impotenza della pubblica amministrazione. Se un'amministrazione approva una legge nel 1998 per regolare il mercato dell'affitto, la legge n. 431, e adotta un provvedimento di proroga che viene poi riproposto per sei anni consecutivi per alcune tipologie contrattuali, nonostante il richiamo della Corte costituzionale, è evidente che siamo di fronte ad un'anomalia. Un'amministrazione e un Parlamento che operano in questo modo hanno una palese difficoltà ad individuare risoluzioni concrete. La Corte costituzionale, già tre anni fa, invitava il Governo a non prorogare in continuazione, perché la proroga non può sostituirsi alla legge; lo strumento della deroga di un provvedimento legislativo in vigore non può che avere un carattere transitorio e limitato nel tempo. Voglio però ricordare che, questa volta, siamo in una condizione del tutto particolare, perché siamo di fronte ad un disegno di legge e non ad un decreto‑legge, a causa della decadenza, nell'ottobre 2006, del decreto-legge predisposto dal Governo a seguito del voto sulla pregiudiziale di costituzionalità da parte del Senato. Quello, se mi è consentito dirlo senza rientrare nella polemica, è un classico esempio di calcolo miope, perché un successo di tattica parlamentare di corto respiro veniva giocato sulla pelle di cittadini bisognosi. Quel voto ha creato un vuoto che ha portato all'esecutività di alcuni sfratti ed impone oggi al Senato di approvare nei tempi più brevi possibili il provvedimento Questo percorso legislativo così irto di difficoltà, insieme con le recenti pronunce della Corte costituzionale sulla materia, hanno imposto al legislatore di avviare un procedimento legislativo innovativo, non limitandosi ad una mera riproposizione del blocco temporale e temporaneo degli sfratti, ma avviando anche una fase di programmazione concertata che provi ad offrire una soluzione ad una tematica così complessa. Voglio provare

Ma la situazione è divenuta difficile anche per l'evolversi di alcune dinamiche economiche: la fuga dei capitali dalla Borsa all'inizio del terzo millennio ha fatto galoppare i prezzi degli immobili, con inevitabili conseguenti lievitazioni degli affitti, che oggi arrivano a richiedere il 40 o anche il 50 per cento del reddito disponibile per le famiglie; le operazioni di cartolarizzazione hanno depauperato il patrimonio immobiliare pubblico; si è nettamente ridotto il fondo sociale per il sostegno alle locazioni; per i giovani si è fatto sempre più difficile l'accesso ai mutui, sia per la selvaggia precarizzazione dei rapporti di lavoro, sia per la nuova stagione di incremento dei tassi di interesse. Tutto questo, in uno con la particolare situazione della proprietà immobiliare che vede una percentuale pari a circa l'80 per cento di cittadini proprietari di abitazione, costituisce un indiscutibile freno alla mobilità territoriale della popolazione.

esposti tra l'altro a fenomeni di selvaggia speculazione e a tragedie come quelle che abbiamo recentemente vissuto a Roma. Occorrerà quindi, dopo l'approvazione di questo provvedimento, lavorare seriamente per realizzare una indispensabile concertazione tra Stato, Regioni, enti locali, sindacati degli inquilini e dei proprietari, perché appare indispensabile una preliminare fase di ricognizione che individui programmi, risorse, leve fiscali, tutti gli strumenti in grado di avviare a soluzione il problema.

come rinnovare nel nuovo *welfare* la cultura stessa dell'intervento pubblico nel settore; come rinnovare gli strumenti di gestione dell'immenso patrimonio di edilizia pubblica e come integrare i programmi di intervento nelle politiche di riqualificazione delle città. Occorre puntare sul recupero e il riuso delle aree urbane e sulla riqualificazione delle periferie, coinvolgendo i privati anche al fine di velocizzare la realizzazione dei piani (sappiamo che dalla elaborazione di un programma di intervento pubblico alla sua concreta realizzazione passano mediamente sette anni). Nessuno, quindi, si illude che questo sia l'ultimo provvedimento in materia di disagio abitativo, ma speriamo che sia l'ultimo che viene adottato senza una seria ricognizione del patrimonio pubblico, delle condizioni di Comuni e Regioni e, soprattutto, senza la disponibilità

del provvedimento legislativo in esame, urgenza legata alla circostanza che il disagio abitativo in forma di sfratti sta oggi interessando centinaia di persone in tutto il Paese

sulla necessità che si riapra in questo Paese una seria politica abitativa: o siamo nelle condizioni, con i tempi che il Parlamento avrà, con le risorse che troveremo, di rimettere al centro delle questioni il problema casa come uno dei diritti esigibili e quindi come una delle priorità che questo Governo e questa maggioranza devono assumere, oppure davvero, come ci ricordava poc'anzi il senatore Piglionica, rischiamo di ritrovarci a rinnovare ogni anno la questione dell'emergenza sfratti con una ritualità assolutamente insopportabile, peraltro anche contrassegnata da appunti severi da parte della Corte costituzionale. Quindi, ritengo che nel disegno di legge questa opportunità sia stata scandita da proposte che, in relazione con i Comuni, con le Regioni e con le parti sociali, possono contraddistinguere i prossimi mesi come i mesi della elaborazione di un piano casa, capace di disegnare il futuro del diritto all'abitazione. Mi pare che queste siano le due condivisioni che siano state rimarcate in questo dibattito. Per questa ragione penso che avremo davanti mesi operativi molto importanti. Tre precisazioni infine al senatore Pastore, perché i suoi appunti sono molto puntuali e credo quindi vadano assolutamente interpretati come tali. Intanto l'ampliamento dell'ambito di applicazione, da lui definita la platea dei Comuni.

da un'esigenza reale che sul territorio del nostro Paese c'è. Lo dico anche perché i senatori e le senatrici sanno che questo provvedimento si riferisce agli sfratti per finita locazione, quindi non tratta la questione più generale degli sfratti, che pure esiste, anche in termini molto forti; quindi, a maggior ragione, essendo un ambito ridotto in termini di applicazione, la richiesta è stata proprio quella che perlomeno l'ambito

relatore, quella corretta mi sembra abbastanza evidente: i figli a carico sono un'altra declinazione di un disagio familiare che però risponde al criterio di famiglie con un reddito di 27.000 euro e che non abbiano altre abitazioni. che non abbiano altre abitazioni. Non so se è un'interpretazione o è un'interpretazione autentica. A me pare che questo sia l'elemento interpretativo

che propone un'altra questione che riguarda le botteghe storiche, che in forma di emendamento ovviamente non può essere accolta, ma ove il senatore volesse trasformarlo in un ordine del giorno, personalmente credo che si potrebbe accoglierlo perché risponde a un problema vero. È chiaro che con l'articolo 7 si è inteso determinare un equilibrio possibile o un equilibrio migliore e che certamente, parlando di equilibri, si è sempre nel campo della virtualità e dell'approssimazione tra un diritto e un valore, come quello della proprietà, e un diritto e un grande valore, come quello della collettività, per non vedere disperso un patrimonio straordinario, quello dei teatri, che nel Paese è seriamente a rischio.

ma è stato pensato (è stato anche oggetto di una lunga discussione nella precedente istruttoria, quando si parlava del decreto-legge n. 261 del 2006) proprio come elemento

Penso che il disegno di legge in esame non risolva il problema dell'abitazione e della casa del nostro Paese. I dati che personalmente ho fornito nella relazione evidenziano una situazione così pesante, così drammatica,

Debbo però comunicarvi che, a causa del protrarsi della discussione alla Camera dei deputati, l'informativa del Ministro non potrà avvenire prima di venti minuti.

Onorevoli colleghi, ringrazio il Ministro dell'interno per aver accolto senza esitazione l'invito a venire a riferire all'Assemblea sui gravissimi fatti di Catania. Sono sicuro di interpretare il sentimento di tutto il Senato nel rendere omaggio all'ispettore di Polizia Filippo Raciti ucciso quel tragico venerdì sera. A sua moglie, ai suoi figli, ai familiari va la nostra sincera vicinanza e la commossa partecipazione ad un lutto tanto grave quanto incredibile. Alla signora Marisa Raciti rivolgo poi un sentito ringraziamento per le nobili parole pronunciate ieri alla cerimonia funebre. Ancora una volta una giovane vita è stata stroncata in modo assurdo e insensato durante una partita di calcio. La morte, a trentotto anni, di Filippo Raciti, mentre svolgeva il suo lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico, lascia sgomenti. Ancora una volta una partita di calcio che, come ogni manifestazione sportiva, dovrebbe essere improntata ai valori della lealtà, della correttezza, del rispetto reciproco, dentro e fuori il campo da gioco, si è trasformata in un episodio guerriglia urbana che dei criminali hanno condotto ad un epilogo tragico. Ancora una volta si torna a discutere su come prevenire e reprimere simili manifestazioni di violenza. Ascolteremo le misure che il Governo intende adottare, con urgenza, per raggiungere questi obiettivi. Auspico una forte condivisione in Parlamento della strategia per sconfiggere questa piaga della violenza dentro e fuori dagli stadi, piaga sulle cui cause remote è giusto interrogarsi ma senza mai cedere ad atteggiamenti giustificazionisti. Esprimo poi un apprezzamento per le prime decisioni assunte dalle autorità del calcio, nella speranza che il desiderio espresso da più parti di fermezza contro le degenerazioni, di rigore e restituzione del mondo del calcio ad una dimensione di serenità e di pulizia permanga e superi gli ostacoli frapposti dai tanti interessi che possono condizionarlo. Ribadisco la solidarietà del Senato della Repubblica alle forze dell'ordine, che ancora una volta hanno pagato a caro prezzo il compito di tutelare tutti noi e garantire la sicurezza delle nostre città. Alle forze di polizia, attraverso il Ministro dell'interno, vogliamo far giungere anche la nostra gratitudine per l'impegno che svolgono quotidianamente a difesa della legalità e la ferma condanna per le scritte odiose ed inammissibili apparse nei giorni scorsi in alcune città. La nostra comune speranza è che il sacrificio di un fedele servitore dello Stato non risulti vano, ma aiuti la società a recuperare appieno i valori autentici dello sport e della cultura della legalità. **Comunicazioni del Ministro dell'interno sui tragici

si percepisce in fatti di questa natura. Si colgono le radici specifiche di una violenza che si viene organizzando, che sono a Catania diverse da quelle di Napoli e sono a Napoli diverse da quelle di Bergamo e quindi un segnale di attenzione, di interventi, di responsabilità per la violenza stessa che sono volta a volta diverse. Allo stesso modo, però, dai fatti si coglie una perversa - non saprei come altro definirla - capacità ormai dell'organizzazione del calcio in tanti suoi ingredienti, come catalizzatore amplificatore di questa violenza, ancorché diversamente formata in diversi luoghi. Di qui il senso di una riflessione, di un pronto intervento che deve riguardare non soltanto la città in cui i fatti sono accaduti, ma l'insieme del calcio. La partita Catania-Palermo era prevista dal calendario ufficiale della Lega calcio per il 4 febbraio, cioè domenica ma da tempo destava forti preoccupazioni sia per la rivalità tra le due tifoserie, entrambe della medesima Regione, sia per la concomitanza della data del 4 febbraio con i festeggiamenti per Sant'Agata, che nella tradizione di Catania, come è noto, vanno al di là del fatto religioso e coinvolgono, in un insieme di cortei, di processioni e quant'altro, l'intera popolazione. Quindi si erano tenute già diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dalle quali era emersa l'opportunità di rinviare la partita ad una data diversa e anche la società Catania calcio ha riferito al Prefetto di aver reiteratamente chiesto alla Lega calcio lo spostamento dell'incontro, senza ottenere risposta. Della vicenda si è occupato anche l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, presieduto da un alto dirigente del Dipartimento di pubblica sicurezza, nel quale sono presenti altre amministrazioni, a partire dal Ministro per le attività sportive, e i rappresentanti del mondo calcio. È un organismo che ora ci servirà molto, anche per il futuro, compie un monitoraggio complessivo della situazione della sicurezza e che valuta anche le singole situazioni. L'Osservatorio concludeva, il 25 gennaio, che nelle condizioni date il livello di rischio di quell'incontro era pari al livello 3 - che corrisponde al rosso di altre nomenclature, cioè il massimo livello - e quindi proponeva di differire ad altra data l'incontro.

il venerdì, però alle ore 15. Sottolineo l'importanza dell'ora perché il livello di sicurezza e di rischio, come è facilmente comprensibile, è ritenuto più elevato, al massimo della sua possibile elevatezza, nelle ore notturne e lo è di meno se la partita si svolge nelle ore diurne. Nella riunione successiva del Comitato provinciale entra, finalmente con una sua presa di posizione scritta, la Lega calcio, la quale, in relazione all'impossibilità, di cui prende atto, di far svolgere l'incontro o il sabato o la domenica, tuttavia rifiuta l'ipotesi del differimento e insiste perché l'incontro abbia luogo il venerdì, sottolineando che il calendario successivo è stracolmo, che non ci sono altre date che rinviare a date successive provocherebbe lo scombinamento del campionato. Quindi, si propone venerdì 2 naturalmente alle ore 18, perché ci sono i contratti televisivi e perché - notano le autorità locali - in una giornata lavorativa alle ore 15 non permette a chi stia ancora lavorando di andare allo stadio. Alla fine, in questo contesto, viene disposto dal Prefetto che la partita abbia luogo il venerdì 2 febbraio alle ore 18. A quel punto, inizia la vicenda dell'assembramento della tifoseria locale all'interno e all'esterno dello stadio. Ci sono 20.000 persone. La tifoseria palermitana è in viaggio - per circostanze accidentali, incredibilmente lento - da Palermo. Partono in ritardo i pullman accompagnati dalle forze dell'ordine,

che raggiungono Catania molto più tardi dell'inizio della partita e i tifosi entrano nello stadio alle ore 19,15, quindi a secondo tempo già iniziato. A quel punto i tifosi catanesi tentano un'aggressione nei confronti dei subentranti tifosi palermitani. Ci sono lanci di pietre e di altri corpi contundenti tra tra l'interno e l'esterno dello stadio, perché una parte dei tifosi è rimasta fuori dallo stadio. Le forze di polizia ricorrono a lacrimogeni e riescono, grazie a questo e al loro intervento, ad evitare che le due tifoserie entrino a contatto diretto l'una con l'altra. Ai lacrimogeni della polizia si sommano i fumogeni tirati dai tifosi. Si crea quel nebbione tipico di determinate situazioni. L'arbitro sospende la partita, che rimane ferma per quasi mezz'ora. Poi si sollevano i fumi e la partita riprende, arriva alla sua conclusione, ma intanto fuori prende fuoco l'azione nei confronti della Polizia e i tifosi del Palermo rimangono sotto assedio chiusi dentro lo stadio. La Polizia si trova a lottare in un clima di autentica guerriglia, che credo molti di voi abbiano visto in televisione grazie all'emittente che si è collegata in diretta con Catania nella tarda serata di venerdì. Da una parte, quindi, la guerriglia; dall'altra, l'esigenza di coprire i tifosi del Palermo, che rimarranno a lungo prigionieri dello stadio, ma senza conseguenze fisiche

del quale inizialmente apprendiamo che, davanti al fumo di qualcosa di fumogeno, scende dalla macchina su cui sta lavorando, ne viene colpito (perché in realtà è una bomba carta che esplode) e viene portato in rianimazione. Le agenzie di stampa dicono che è morto, ma in realtà non è vero, perché egli è ancora vivo e morirà un'ora dopo stato portato all'ospedale. In seguito, apprenderemo che è deceduto a causa di un trauma addominale e fratture multiple del fegato compatibili con un corpo contundente di importante adeguatezza lesiva. Quindi, non è stata la bomba carta. Quest'ultima, evidentemente, ha provocato un trauma finale, in parte cardiaco e in parte emotivo, immagino, ma in realtà il nostro ispettore, che era stato colpito prima da un corpo contundente (immagino un masso; non so se fosse una spranga, ma sembrerebbe piuttosto un masso), ha continuato a prestare servizio nonostante ciò e, a seguito dell'esplosione della bomba carta,

iniziano gli arresti, vengono arrestate 33 persone fino a ieri sera, più il custode dello stadio ieri (e arriviamo a 34).

dell'interno*. Sono tenuto a dare un'informativa al Senato. In questo momento sto informando il Senato della Repubblica che non ne è mai stato informato. Sono lieto che lei sia qui e se non è interessato mi lasci per ora concludere. GRAMAZIO *(AN)*. Se sto dell'interno*. Allora non lo posso dire; lei mi ha messo in condizioni d'interloquire con lei, altri non lo hanno fatto. La procura della Repubblica di Catania, a seguito delle perquisizioni effettuate e delle prime indagini, è anche arrivata a sottolineare che, allo stato, non possa escludersi che i gravi disordini siano stati espressione di un preordinato attacco che ha avuto come unico e reale obiettivo le forze di polizia, nei confronti delle quali, peraltro, già nel recente passato si sono dovute registrare reiterate manifestazioni di violenza verbale e fisica. Il racconto dei fatti, larghissimamente noti, si conclude qui, perché proprio la sottolineatura della procura ci fa capire che qui c'è qualcosa che riguarda il rapporto tra violenza, utilizzazione politica della violenza e ostilità nei confronti delle forze di polizia. C'è qualcosa su cui dobbiamo lavorare per capire da dove viene. Certo, si rischia in buona parte di fare quella che, con parola ingiustamente sprezzante nei confronti della sociologia, si chiama la sociologia della criminalità. Non condivido lo sprezzo verso la sociologia, ma mi rendo conto che in questo caso non basta, anche se non la si può ignorare: non si può ignorare quello che mi diceva il Prefetto ieri, di quanti giovani dei quartieri degradati della periferia di Catania, avendo il padre in carcere, o appena uscito o in procinto di andarci, considerano istintivamente il poliziotto il loro nemico, il nemico della loro famiglia. STORACE

Quindi, vi sono ragioni che attengono ad una vita malata della città, ad una identità difficilmente trovata dai giovani, ad un rapporto nel quale essi si trovano con organizzazioni ultrà che li inducono ad associarsi, ad aggregarsi, a farsi valere attraverso questo modo di esprimere un odio quale, come è stato notato, il bersaglio tende ad essere sempre meno la tifoseria avversaria, anche se la tifoseria avversaria è l'occasione per farlo emergere. Quindi - come dicevo all'inizio - siamo di fronte a un problema generale del quale ci dobbiamo occupare, che vedo emergere in una città quale Napoli nella facilità con la quale azioni di per sé criminose, come lo scippo e il piccolo furto, si accompagnano a una dose crescente di violenza nei confronti delle persone che ne sono vittime: in fondo, è una violenza

contesto, legati alle dimensioni del fenomeno calcistico e alla sua portata. Sarebbe ingiusto dire che è lo sport in quanto tale che se li porta dietro.

forse sociologicamente rappresentano segmenti di società in parte diversi da quell'insiemistica più ampia che è sugli spalti di una partita di calcio, ma certamente lì non vi sono incidenti. Alcune specificità del sistema calcio

Ho già riferito alla Camera dei deputati che nella scorsa legislatura, in particolare, sono state adottate misure che portano il nome del mio predecessore qui presente, il senatore Pisanu,

Certo è che oggi ci troviamo in una situazione nella quale l'adempimento nei confronti di quegli *standard* è stato parziale. Alcune fenomenologie regolate da quelle misure - mi riferisco, in particolare, alla vendita in blocco dei biglietti alle tifoserie della squadra ospite e all'organizzazione collettiva dei viaggi non hanno funzionato come ci si aspettava quali riduttori della violenza. Al contrario, il viaggio organizzato ha aumentato, purtroppo, le occasioni di rischio negli autogrill

forse nella stessa inadempienza che hanno subìto, hanno risentito del fatto che il destino complessivo degli impianti sportivi, il loro essere tra le società gestrici e enti territoriali di Governo proprietari, ha creato disincentivi a una responsabilizzazione complessiva delle società sulla loro utilizzazione. Dunque, noi partiamo da queste constatazioni; partiamo oggi dalla necessità di rafforzare e, dove necessario, raddrizzare, come sostenuto ieri parlando agli interlocutori dello sport, le misure già adottate e di collocarle in un orizzonte più ampio (al quale però dobbiamo lavorare subito) che porti a impianti sportivi affidati alle società, dei quali le società assumano finanziariamente e gestionalmente la responsabilità, con la possibilità di farne dei luoghi polifunzionali, creando nelle società forti incentivi a difenderli nelle attività che vi si svolgono.

io non ci mando più i poliziotti nella situazione in cui si trovano», abbiamo preso una decisione che deve essere confermata nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sento che ciò è necessario per tutti: per le famiglie che vanno allo stadio, per la tranquillità di chi

si trovano a rischiare tutte le domeniche per consentire che questo gioco sia un gioco. Non è possibile che a una partita di calcio si debbano dedicare 1.500 uomini. uomini. È chiaro che si è determinata una situazione non normale, se si arriva a quel punto. Ricordavo poco fa alla Camera che

due ragazzi accanto, un bambino e una ragazzina di 15 anni. Una donna di straordinaria forza aveva perso il marito davanti allo stadio

Prima di lei aveva parlato un poliziotto, commosso come tutti i suoi colleghi. Vedevo questi uomini robusti con le lacrime, che silenziosamente uscivano dai loro occhi. Egli, dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato a loro rivolto, ha chiesto che gli si dicesse: noi ci crediamo ancora.

A me spiace quando qualcosa viene comunicata alla stampa prima che alle Camere ma, quando si convoca una riunione a Palazzo Chigi, bisogna informarne la stampa subito dopo. E lo abbiamo fatto prima che potessi venire a dirlo qui, a voi. Fondamentalmente, questo è un progetto

sulla base dell'adempimento rispetto agli *standard* Pisanu, che sono comunque essenziali, di arrivare a ciò che è stato quasi unanimemente proposto in Italia,

il che non sarebbe possibile se non ci fosse tutta quell'opera di prefiltraggio e selezione che è essenziale per ridurre fortemente il rischio dell'incidente all'interno dello stadio. Allora, l'adeguamento deve avvenire e se non avviene gli stadi non hanno il pubblico. Non abbiamo alcuna ragione di tenere il campionato fermo fino a quando tutti gli stadi non saranno adeguati, ma in quelli non adeguati, se si vuole giocare, si gioca a porte chiuse. So benissimo che gli incidenti possono avvenire anche fuori dallo stadio, ma state pur tranquilli che se la partita è a porte chiuse è difficile che attorno allo stadio ci sia lo stesso tipo di assembramento che c'è quando la partita è a porte aperte. Questo mi pare assolutamente ovvio e le società devono capirlo.

al punto di avere stadi che certificano come propria capienza 9.999 spettatori in presenza di una soglia minima che quei decreti fissavano a 10.000, capisco che, a questo punto, qualcosa bisogna fare, perché non posso contare su queste società *rebus* *sic stantibus* per avere l'ottemperanza, avendo già esse deciso l'inottemperanza,

Ancora dobbiamo definire il numero, ma verrà abbassata in modo che il «9.999» ricada comunque nei decreti Pisanu; poi vedremo, ci potranno essere requisiti di minore portata per gli stadi più piccoli. Ci dovrà essere l'ottemperanza comunque: le risorse dovranno essere trovate. Se non vengono trovate, lo stadio continuerà ad essere utilizzato a porte chiuse. Ci dovrà essere, naturalmente, una maggiore severità, e non tanto delle norme. Un collega deputato notava, con finezza latinista, che diverse di queste norme finiscono per essere *minus* *quam perfectae* in quanto c'è il precetto, ma non la sanzione, ovvero quando la sanzione è scritta è soltanto apparente. I reati da stadio non sono reati minori e questo lo deve capire anche chi se ne occupa in sede giudiziaria:

C'è una proporzionalità complessiva nel sistema penale, per cui l'entità della pena è già adeguata. Casomai, a noi serve la quasi-flagranza a quarantotto ore, e questo intendiamo riproporlo, riferita agli accertamenti da fare sulla base delle rilevazioni del videocontrollo *in* *loco* e a quel momento, non sulla base di elementi successivi che, come tali, in realtà renderebbero la quasi-flagranza una cattura mascherata. No! Si deve sempre trattare di un arresto determinato dalla visione del videocontrollo iniziale. Ma ci vuole il tempo necessario a questo fine. Occorre che le sanzioni siano praticate e che quindi siano comminate ed effettive. Occorre che il divieto di frequentare gli stadi sia reso

ha reso impossibile estenderlo ai minori. D'altra parte, troverei aberrante portare l'imputabilità dei minori a 12 anni per potervi applicare questa misura. Non lo farei mai. Ma se questa diventa misura di prevenzione rispetto alla quale il comportamento violento allo stadio è un indice di pericolosità e non una fatto-reato, la misura può essere comminata anche al minore,

che li impegni effettivamente e visibilmente nelle ore durante le quali si svolge la partita. Non dobbiamo ridere davanti a queste circostanze perché queste circostanze perché corrispondono in campo automobilistico al togliere la patente, l'unica iniziativa che scoraggia veramente dall'eccesso di velocità. Altre sanzioni non hanno il medesimo effetto. E non vi è nulla di autoritariamente barbarico nell'imporre sanzioni di questa natura, in particolare ai giovani, che dobbiamo educare meglio ma che dobbiamo anche saper punire quando è il momento di punire comportamenti che, altrimenti, diventano la norma quando la norma essi non possono essere. Dobbiamo cambiare per le tifoserie.

a rischio, rappresentati dai viaggi delle tifoserie e la loro presenza «in pacco». E questo è propedeutico ad un sistema nel quale i rapporti collusivi tra le società e le tifoserie debbono finire. La storia dei biglietti è uno dei modi attraverso i quali le collusioni si mantengono. Non a caso venne giustamente introdotto il biglietto nominativo, proprio per evitare che le tifoserie disponessero liberamente dei biglietti e li gestissero come volevano.

dell'odio razzista, dell'odio contro il presidente della Lazio che li ha privati di risorse, di cui prima si potevano comodamente avvalere, di una ostilità che non è neanche l'amplificazione dell'antagonismo sportivo, ma che nulla ha a che vedere con l'antagonismo sportivo. E bisognerà anche occuparsi di coloro che in questo fanno gli eccitatori e gli istigatori all'odio. È un'idea alla quale sta lavorando Giovanna Melandri, va attuata con il massimo di attenzione, ma sono troppe le radio e le televisioni locali che fanno eccitazione e istigazione continua alla violenza e all'ostilità.

(che sarebbe per ciò stesso censorio), che si occupi di segnalare e stigmatizzare queste forme di istigazione. Insomma, lo sport è agonismo e anche antagonismo, e tale non può non essere, ma che lo sport generi il nemico contro il quale si esercita violenza questa è cosa alla quale dobbiamo porre rimedio. Mi fermo qui, perché ho già parlato anche troppo. Ci saranno altre misure. È importante che partano entrambe le cose. Credo che convincere oggi le società a farsi carico degli adempimenti cui non hanno ancora provveduto, senza dare la prospettiva che lo stadio sarà loro,

colleghi, che nel 1995 si trovò a sospendere il campionato dopo che c'era stato un morto; eccoci qui, dodici anni dopo, c'è stato un altro morto e sospendiamo il campionato. Impariamo dalle esperienze, capitalizziamo la parte positiva che queste ci hanno dato e andiamo oltre, in modo da riuscire a liberarci di questo cancro (permettetemi di dirlo, il modello inglese è molto citato), senza bisogno di avere 88 morti come in Inghilterra per arrivare a un drastico cambio di registro. Credo che l'immagine di quell'ispettore, di sua moglie, di sua figlia e di quegli altri agenti che ho visto ieri dovrebbe essere un monito sufficiente per noi per intervenire per il mondo del calcio per cambiare. Lo spettacolo non può continuare a questo prezzo. Ci saranno grandi interessi economici nel calcio, entrate fiscali dipenderanno dallo svolgimento delle partite, colossali partite di diritti televisivi sono in ballo quando si parla del calcio, ma, Santo Signore, manteniamo le proporzioni: non si può morire per questo, quand'anche si tratti dello sport più gigantesco e più lucrativo del mondo.

in servizio, una persona perbene nel lavoro a nella vita. Ci inchiniamo di fronte a questo eroe, vittima di una violenza inutile e ingiusta che lo ha visto cadere, e rendiamo omaggio al dolore della sua famiglia, ora priva di un padre e di un marito. Balza evidente dalle affermazioni del signor Ministro dell'interno che ci sia stata una grave sottovalutazione del contesto complessivo, della concomitante festività in onore di Sant'Agata, da parte della Lega calcio. Oggi il nostro dibattito deve servire a confermare, o se volete a rafforzare, la linea del Governo e le decisioni prese in sede di incontro tra il Governo e i massimi vertici dello sport (il CONI e la Federcalcio) che faranno parte di un pacchetto di misure legislative annunciate, che verranno assunte dal Consiglio dei ministri straordinario di domani. Preso atto che in Italia ci sono molti stadi non a norma e che ci sono già norme vigenti che prevedono che questi luoghi deputati a ospitare eventi sportivi debbano essere adeguati a *standard* di sicurezza più elevati, bisogna, una volta per tutte, fare rispettare le norme già esistenti e, se necessario, bisogna anche aggiornare e migliorare quelle norme alle nuove esigenze. Come ha giustamente rilevato il Ministro dell'interno, a questo punto l'ordine pubblico diventa la prima priorità, abbattendo remore, pigrizie, superficialità, negligenze, connivenze, l'ultima grave, senza scampo, quella del custode dello stadio, basista di facinorosi e fornitore di attrezzature contundenti. Il primo punto è quindi che non si gioca con il pubblico in stadi che non rispondono alle normative vigenti; si deve giocare solo negli stadi a norma. Le norme vanno anche migliorate e quindi va eliminata la canalizzazione delle tifoserie che ha portato, tra l'altro, a scontri incivili tra tifosi. Bisogna insomma dare meno potere alla tifoseria organizzata, i cui capi spesso finiscono per condizionare in modo negativo il comportamento dei ragazzi più giovani. A Catania, come in molta parte del Mezzogiorno, siamo poi di fronte a giovani che nella maggior parte dei casi non vedono un futuro; la speranza di uscire dal degrado morale o dall'emarginazione sociale in cui vivono per loro è debolissima. Il divieto di frequentare uno stadio deve poter diventare una misura di prevenzione in presenza di soggetti che abbiano già dimostrato di essere pericolosi e deve essere adottato anche se non si è in presenza di una precedente commissione di reato. Così come condividiamo l'estensione della flagranza di reato a quarantotto ore che può consentire l'individuazione dei responsabili di reato o comportamenti illeciti all'interno o nei dintorni dello stadio. Il lavoro delle forze di polizia è un lavoro straordinario; eventi sportivi, come le partite di calcio, tolgono molti uomini ad altri compiti di pubblica sicurezza nelle città. Le società sportive devono quindi prendersi le proprie responsabilità e devono investire nella sicurezza ammodernando gli stadi, ove di proprietà; non è possibile porre all'esclusivo onere dello Stato e della forza pubblica il problema della sicurezza legato alle partite di calcio. Crediamo che il Governo e gli enti sportivi abbiano individuato le misure adeguate a risolvere una volta per tutte questa emergenza. La Sicilia subisce un'altra brutta mazzata per colpa di un branco di assatanati, di delinquenti senza scrupoli, contagiati da un contesto paramafioso fatto di attacchi alle forze dell'ordine, di insulti e di illegalità di ogni tipo; un contesto che può rappresentare la precondizione per preparare il terreno per scorribande più sanguinarie contro lo Stato e i suoi presidii preposti all'affermazione della legalità e della sicurezza. A ciò dobbiamo e possiamo ribellarci. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato con estrema attenzione la sua relazione. Anche quando ho avuto la tentazione di interromperla perché la sua ricostruzione stava inclinandosi verso un'interpretazione troppo localizzata della vicenda, ho fermato l'istinto e ho atteso che concludesse per intero il ragionamento. ragionamento. Lei ha cercato - la ringrazio per questo - di inserire la vicenda disgraziata, che ha riguardato la mia città qualche giorno fa, all'interno di un'analisi di contesto più ampia che trova in questa occasione una sorta di emblematica vicenda che concerne il disagio di una generazione giovane e che attraversa complessivamente questo Paese nelle più diverse condizioni economiche, sociali e civili. Cosa tiene insieme le scritte di odio per la Polizia che compaiono sui muri di Bologna, di Livorno, di Palermo e di Roma, questo disvalore così enorme, questo disconoscere i segni minimi della nostra convivenza civile questa contestazione brutale dei princìpi di autorità? La ricostruzione della vicenda apre uno squarcio drammatico su questa generazione di giovani e sulle loro inquietudini profonde. Tra la ricerca di un protagonismo, anche fortemente identitario, com'è quello con cui si organizzano gli ultras e tutte le organizzazioni con queste caratteristiche, e l'odio per le forze dell'ordine vi è uno spazio drammatico davvero pericoloso per la crescita di questa nostra società. Il rapporto con il calcio, colleghi, appare quasi accidentale. L'evento agonistico in quanto tale non c'entra nulla, se non come occasione strumentale del potersi confrontare o con l'esercito avversario - l'altra tifoseria - o, quando questo ti è impedito, con le forze dell'ordine, soprattutto quando esse sono efficienti, determinate e quindi, in qualche modo, esaltano il conflitto di questi facinorosi. In tal senso, voglio esprimere

all'ispettore capo Raciti, mio concittadino, che anche nelle modalità della sua morte rende evidente il senso di sacrificio di dedizione: pur colpito da un corpo contundente con danni gravissimi, che ne hanno determinato la morte - era, dunque, falsa la pista della bomba carta -, ha continuato ad operare sino ad accasciarsi con una dedizione straordinaria. Non credo di essere l'unico, perché molti altri si allineeranno a questa proposta, a ritenere che, proprio per le modalità che hanno superato l'ordine normale di comportamento di un fedele servitore dello Stato, quest'uomo vada

umano e politico che dovrebbe richiamare a responsabilità chi volesse restare nel torbido di questa vicenda per inserirvi elementi estranei

Evitiamo, però, se non abbiamo elementi certi, di confondere le acque, di innestare in questa vicenda elementi che ne sono estranei. Per

Evitiamo però i polveroni, evitiamo di giocare le partite della politica squallida, trascinando nel fango istituzioni e responsabilità estranee. Individuiamo, invece,

seguito di questa vicenda assumono cogenza e vigore. Capisco anche l'orizzonte complessivo che riguarda il pianeta calcio.

Occorre capire dov'è il nocciolo delle responsabilità, dove vi sono le solidarietà, quali i luoghi fisici e le relazioni che consentono a questo sistema di degenerare nella violenza e nell'aggressione alle autorità e alle forze di polizia che sono presidio di garanzia democratica. Questo riferimento deve però appartenere a tutto il Parlamento. Provo grande fastidio quando miei colleghi parlamentari, nella libera manifestazione del loro pensiero, continuano a coltivare

Non è strumentale ricordare che se c'è stato un momento in cui in questo Paese è ricominciata un'opera di delegittimazione e di contestazione delle forze dell'ordine e di coloro che garantiscono l'ordine pubblico, in particolare quel momento è da

evocato una tragedia che nulla ha a che fare con gli episodi di Catania c'era il nome di Carlo Giuliani. Si mischiano in queste vicende troppe cose. Facciamo chiarezza, allora, e soprattutto evitiamo

«Vorrei che il sacrificio di mio marito servisse a qualcosa». Con queste parole,

una fermezza e una umanità che sono un esempio per tutti. Signor Ministro, ieri mattina nella Cattedrale di Catania c'era un'atmosfera un po' surreale: la scelta di continuare i festeggiamenti di Sant'Agata, sia pur in forma misurata,

accoglie il giorno della festa di Sant'Agata, stridevano un po' con quella bara poggiata per terra, davanti all'altare. Ma la città ha dato un segno forte di indignazione e di risveglio; la chiesa era stracolma di migliaia di persone, così come le strade e piazza Duomo. correttamente, signor Ministro, come lei ha fatto, quanto è accaduto. Vi è certamente una componente di violenza calcistica nella guerriglia urbana di venerdì sera nella mia città, a Catania,

la scelta di non consentire più l'acquisto in blocco di biglietti per la tifoseria. Non è immaginabile che dal 1° gennaio ad oggi oltre 100.000 appartenenti alle forze di polizia siano stati impegnati a scortare le tifoserie in trasferta:

l'impostazione del Governo nei confronti dell'azione di medio periodo tendente a responsabilizzare le società di calcio. certamente pressioni in quest'Aula del Parlamento, come alla Camera, come al Governo, da parte di quel mondo che ruota intorno al calcio e che vorrebbe che tutto rimanesse come è stato fino a questo momento. Credo che il monito della signora Raciti debba risuonare nelle orecchie di ciascuno di noi: linea dura dal punto di vista repressivo, oggi, e un'azione di responsabilizzazione. Non possiamo far finta che nulla sia accaduto. *(Applausi dai

Il tono di oggi ci fa capire quanto sia stata sentita la presenza del Ministro, che ringraziamo innanzitutto per averlo avuto ieri a Catania. ci dispiace che il ministro Melandri sia andata via, ma la ringraziamo veramente perché ha dato testimonianza di come lo Stato voglia, con forza, essere vicinoalla famiglia Raciti, una famiglia alla quale siamo vicini e alla quale Catania è vicina. Una Catania che, Presidente, Ministro, viene in questi giorni dipinta come una città che ha bisogno di un intervento in più,

una città che ha rialzato la testa ormai da anni, che non è un caso nazionale. Quanto detto dal prefetto è vero nella misura in cui è vero anche a Bologna, a Bergamo, a Venezia, a Noto, a Ragusa o maggiormente a Napoli: il degrado delle periferie, la disaffezione alla scuola, la criminalità. Catania non è un caso. Catania è quella città che ha superato i 100 morti l'anno precedenti all'amministrazione Scapagnini, con un tasso di criminalità fortemente ridotto dal punto di vista della mafiosità. Catania è quella città che ha avuto finalmente un'amministrazione non toccata da gravi reati attinenti alla pubblica amministrazione o ad essa vicina. Catania è quella città che ha riscoperto al posto delle baracche a San Giorgio le scuole,

l'ospedale San Marco, il poliambulatorio con 5.000 visite l'anno. Lei, presidente Marini, conosce la città di Catania e le sarei grato della sua attenzione. Catania è quella città nella quale la disoccupazione è scesa del 6 per cento da quando è amministrata dal professor Scapagnini e Scapagnini e che, da quando è amministrata dal centro-destra, riesce ad avere all'interno del suo centro infrastrutture totalmente cambiate, restituite al barocco e ai turisti che vengono nella nostra città, offesa da dei criminali che sono paragonabili a quelli filocomunisti della tribuna tribuna di Livorno. A Catania possono essere di segno diverso, ma quelle tifoserie sono ambedue da condannare e spero che il Ministro lo faccia, non appena avrà un minuto dopo aver terminato il suo colloquio*.

non perché appartiene a questo Governo, ma perché è lei. Come possiamo, infatti, avere fiducia in un Governo nel quale la divisa dopo il G8 è vista come un nemico?

Ma possiamo avere fiducia in un Governo nel quale c'è gente che ha avallato ed è stata vicina alle manifestazioni di piazza nelle quali si sono bruciate le divise di soldati americani e italiani, gridando «Dieci, cento, mille Nassirya»? E speriamo che un'aula,

frequenza, torna ad insanguinare i nostri stadi impone, dopo l'ultima intollerabile prova di forza, una riflessione seria e profonda su varie questioni. Comincio da quella che solo apparentemente è la cornice formale del problema, e cioè l'ennesima grottesca passerella di dichiarazioni inopportune con cui, all'indomani della morte dell'ispettore capo Raciti, è stato violato quello spazio prezioso che una composta liturgia laica del dolore imporrebbe. Per il mondo della politica il mio pensiero sdegnato corre ad un parlamentare tra i più extraparlamentari della nostra maggioranza, ha parlato di una pretesa mancanza di addestramento delle nostre forze dell'ordine, chiedendo di poterle identificare con dei numeri sull'elmetto, mentre tutti noi ci interroghiamo su come identificare gli assassini che siedono, impuniti ed occulti, nelle curve degli stadi accanto ai comuni tifosi. Complimenti all'onorevole Caruso per la sua squisita sensibilità ed anche per la sua capacità di essere sempre e comunque controcorrente rispetto agli indirizzi generali del Governo. Voci stonate provengono anche dal professionismo sportivo. La posizione di Matarrese ha puntato unicamente e cinicamente sulla necessità di non fermare il grande *business*. Il mondo dei *club*, degli *sponsor*, dei dirigenti sportivi ha detto la sua: lo *show* deve continuare a qualsiasi costo. Basterebbe solo questo a farci capire quanto igienica sarebbe una chiusura temporanea degli stadi e non solo per allestire le necessarie deterrenze contro il il profilarsi di una nuova razza di belve da stadio. In questa prospettiva la violenza, il vandalismo, gli scenari di guerriglia urbana, le scritte infamanti contro il servitore dello Stato lasciato sul terreno a Catania a Catania non sono più il mezzo, ma il fine ovvero la manifestazione estrema di un ribellismo a geometria variabile e di una determinata cultura del nemico che ora compatta l'eterogeneo branco degli ultras contro il più assoluto e primordiale dei nemici: l'ordine e dunque lo Stato. In tale prospettiva desidero confermare piena solidarietà al ministro Amato. Parallelamente devo prendere le distanze da chi nell'opposizione, ma anche nella maggioranza giudica pretestuosamente inapplicabile alla nostra realtà il cosiddetto modello inglese per prevenire e punire attraverso l'inasprimento delle pene. Riformiamo sul serio il nostro calcio, chiudiamo gli stadi non in regola finché ovunque, da Torino a Palermo, non si chiude il cerchio della deterrenza previsto dalla legge vigente e mai concretamente applicato. I biglietti, che i controlli *ex post* operati a Catania hanno rivelato intestati a Osama Bin Laden o Ludovico il Moro, sono la prova lampante che una vera identificazione agli ingressi di fatto non esiste. Se le disponibilità dei Comuni non bastano a rendere operativo il sistema, allora si privatizzino gli stadi, come propone il ministro Melandri oppure, come suggerirebbe il guardasigilli Mastella, si faccia cassa obbligando i *club* ad investire parte dei diritti televisivi nella sicurezza delle partite. conclusione, il calcio italiano è morto, come titolava amaramente in questi giorni il quotidiano della Santa Sede commentando l'infernale sabba calcistico di Catania. Io, da da inguaribile ottimista qual sono, credo che il nostro calcio sia semplicemente molto, molto, molto malato. Se è guaribile o no saranno i provvedimenti che saranno presi in questi giorni a deciderlo.

che io ritengo incompleta e parziale. Ciò che ha ferito il Paese è stato l'oltraggio alle forze di polizia e una risposta che, a mio parere, è stata debole e timorosa rispetto alle forze impegnate. Il decreto Pisanu è stato inattuato e aggirato. Di chi è la responsabilità? Le responsabilità per i reati da stadio ‑ che lei ha richiamato nella loro pericolosità ‑ devono essere certe. Non vi può essere una sospensione condizionale della pena. Si deve vietare il possesso dei fumogeni, delle bombe carta e degli oggetti contundenti. Il problema, signor Ministro, non è la chiusura degli stadi, bensì la loro apertura; lì si misura la capacità dello Stato di fronteggiare la situazione e accettare la sfida. Quest'ultima potrà essere vinta solo quando lei, signor Ministro (mi dispiace che non ci sia il ministro Melandri), potrà andare allo stadio, la prima domenica di apertura,

Non è questo il momento di fare analisi sociologiche, ma dobbiamo ripristinare nei giovani il concetto di legalità e di rispetto per chi tutela la sicurezza e l'ordine pubblico. questo è il primo punto da portare avanti: il rispetto della tutela della funzione della divisa, di chi muore in divisa. Ciò sarà possibile se le misure che verranno adottate saranno adeguate e tempestive, capaci di rimuovere alla radice i problemi che esplosi a Catania, ma che valgono per tutto il Paese.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, di fronte all'ennesima tragedia è urgente interrogarsi a fondo sul senso della cultura sportiva nel nostro Paese. Ci attendiamo interventi e decisioni severe da parte del Governo, capaci di reprimere la violenza nel calcio. Ma questo non può bastare, non deve bastare, né allo Stato né alle istituzioni. Noi, tutti insieme, abbiamo l'obbligo morale, come rappresentanti del popolo sovrano, di non accontentarci di definire le regole e poi delegare alle forze dell'ordine. Abbiamo il dovere di capire e di comportarci con coerenza. Dobbiamo capire come sia possibile che una giornata di festa e di sport si trasformi in una caccia al poliziotto. Dobbiamo capire come sia possibile che un dirigente sportivo, al termine di una partita di terza categoria, venga picchiato a morte da persone che si definiscono tifosi o addirittura atleti. Cosa produce una spinta omicida tale? Cosa spinge un gruppo di persone a diventare un branco? Non possiamo delegare - come lei ha giustamente anticipato - la comprensione di questo fenomeno solo ai sociologi e all'accademia. Se così facessimo, saremmo condannati all'inefficacia e la nostra azione di legislatori sarebbe compromessa. Infatti, è evidente che la questione della violenza non si limita agli stadi. Quei tornelli sono un confine troppo aleatorio per pensare che il problema sia solo lì dentro. Ce ne dobbiamo rendere conto quando vediamo fenomeni di bullismo nella scuola, quando *gang* di strada usano la violenza come codice di vita, quando siamo costretti a rifugiarci in una definizione vaga come il disagio giovanile. C'è un grande e inesplorato problema sociale di fronte a noi che non possiamo limitare agli stadi, ma che investe tutta Vorrei però che fosse chiaro: questo non è e non deve essere un alibi per chi pensa allo sport solo come a un mercato e non come a una passione. Non è un alibi per quelle società che ritengono legittimo essere conniventi con i tifosi più violenti

È un grande problema che dobbiamo affrontare dentro e fuori dagli stadi, negli stadi e nelle scuole, negli stadi e nelle famiglie, negli stadi e nelle periferie degradate di Catania, Napoli, Bergamo, Milano e di altre città italiane. E' urgente allora coniugare tre elementi: una decisa repressione dei reati, una puntuale prevenzione del fenomeno della violenza e un'azione sociale a largo spettro. Senza tutti questi elementi rischiamo la sconfitta. Avremo modo di approfondire provvedimenti che rafforzino le ragioni dell'ordine pubblico. Sono certo che il Governo interverrà con decisione e rapidità e, in quella sede, come parlamentari, entreremo nei dettagli, parleremo della gestione degli stadi e della responsabilità in capo alle società. Ma oggi, a un giorno dai funerali di Filippo Raciti, è doveroso tributare a questo servitore dello Stato il triste omaggio che si deve a chi muore nell'assolvimento del dovere ed è ancora più doveroso dare una risposta alla sua famiglia. «Che la tua morte induca la società a cambiare», questa è stata la speranza espressa dalla moglie di Raciti ieri al funerale. È questo l'impegno al quale io, e spero tutti noi, dobbiamo sentirci legati: cambiare non solo il calcio e lo sport, ma la società. Per chi, come me, ha fatto del calcio un pezzo della propria vita, questo è il giorno in cui è giusto riaffermare anche il senso e il valore dello sport, quello vero, fatto di passione e fatica, di correttezza e disciplina, di saper vincere e saper perdere, di emozione e di regola. Se la repressione è necessaria e urgente, da sola non basta: serve pensare alla prevenzione come processo in cui siamo tutti impegnati, tutti i giorni. Il primo luogo è, ovviamente, la scuola. Ma come possiamo parlare di cultura sportiva se le strutture sono quelle che conosciamo, se le palestre sono un lusso da scuole del centro? Questo è un terreno su cui sarebbe importante rafforzare l'iniziativa tutti insieme, a cominciare dalla prossima finanziaria. Probabilmente è giusto che ci siano meno società miste inutili e più palestre scolastiche, intese come contenitori culturali, a disposizione degli educatori e dei giovani; tutto ciò per recuperare il senso del limite e del rispetto per se stessi e per gli altri. Ormai la nostra società comincia invece a vivere alimentando sempre più la cultura del nemico, non solo nello sport, ma anche in altri campi. Ma la cultura del nemico ha dentro di sé l'idea della violenza e genera solo odio: il nemico si uccide, non si batte e infatti oggi discutiamo a partire dalla morte di un uomo. Anche questo è un terreno su cui dobbiamo fare di più in termini politici e istituzionali, ma soprattutto culturali e di comportamenti - lasciatemelo dire - con esempi e modelli profondamente diversi. Dopo gli eventi degli ultimi anni, aspettiamo di assistere a una rifondazione innanzitutto morale del calcio. Il cammino è in corso e figure alle quali possiamo affidare con fiducia l'autonomia del pallone, come il commissarrio Pancalli, ci sono e stanno lavorando, ma gli eventi di sabato ci dicono che la strada è ancora lunga, perché oggi, tra le questioni all'ordine del giorno, c'è anche quella della credibilità di un sistema. Un'idea di impunità a tutti i livelli alimenta la violenza, non la frena. O tutti gli attori si sentiranno investiti di questo impegno o dubito che ne verremo a capo. Le società e le strutture federali, innanzitutto, non possono pensare che il calcio sia solo un'industria, ma anche i calciatori e le altre componenti hanno la responsabilità dell'esempio. Certamente - permettetemi l'inciso - dichiarazioni come quelle di Matarrese di ieri non aiutano a dare del calcio un'immagina diversa e responsabile. L'importanza assunta negli anni dal mercato, la trasformazione dei *club* in società a scopo di lucro, il dominio delle *pay* TV sugli orari delle partite, un uso distorto dei *media* locali hanno cambiato il volto dell'intero sistema sistema calcio. Oggi il nuovo calcio deve assumersi le proprie responsabilità fino in fondo. Con la legge sui diritti TV stiamo compiendo i primi passi per un'inversione di tendenza, ma anche dal punto di vista della legislazione la strada è ancora lunga. Oltre a tutto ciò servono interventi puntuali. Mi permetto di citare solo tre esempi. Il primo è che non è accettabile che ci sia nel nostro Paese una maggioranza di campi di serie A che ancora non rispondono agli *standard* di sicurezza e in cui non siano presenti sistemi di controllo a circuito chiuso con regia unificata. Ciò vuol dire garantire l'impunità dei violenti e probabilmente lasciare strada libera ai male intenzionati. luogo, dobbiamo rafforzare le risorse anche tecnologiche che le forze dell'ordine hanno a disposizione. I rilevatori di identità nei biglietti, i cosiddetti tag RFID, costerebbero venti centesimi a biglietto; con questo strumento, insieme ai biglietti nominativi, è possibile sapere in ogni momento dove si trova ciascuna persona entrata nello stadio. Gli strumenti per rendere i tifosi responsabili delle proprie azioni Inoltre, è necessario costruire un'alleanza con gli sportivi ed i tifosi contro i violenti, che sono e restano una minoranza. Prima le tifoserie si combattevano l'una con l'altra (ricordiamo tutti la morte di Vincenzo Spagnolo a Genova); oggi i violenti attaccano le forze dell'ordine e questo è un fatto drammatico: il nemico è diventata la Polizia, lo Stato. Dobbiamo sapere che stiamo parlando di una minoranza e che avviare un percorso istituzionale di interlocuzione con il tifo organizzato probabilmente ci può consentire di dividere il grano dal loglio, di ricondurre alla marginalità i violenti. Un'azione sociale e culturale a vasto spettro, a partire dalle scuole: un investimento forte anche economico sulla prevenzione; una puntuale repressione dei delitti: questi devono essere i capisaldi della nostra azione complessiva. Voglio ringraziare il Ministro dell'interno per la puntualità e la rapidità con cui è venuto in Parlamento a riferire e, per suo tramite, voglio esprimere la solidarietà alle nostre forze dell'ordine. Il ministro Amato deve sapere che su questo terreno avrà tutto il nostro sostegno; non solo il Ministro dell'interno, ma tutto il Governo perché da tutto l'Esecutivo ci aspettiamo una risposta: dal Ministro della pubblica istruzione a quello dello sport, da quello della giustizia a quello per la famiglia. Dobbiamo sapere

Per quanto riguarda le impostazioni prospettate stamattina, siamo in totale sintonia con il Ministro e con il Governo. Signor Presidente, Ministro dell'interno, colleghi, a nome del Gruppo Lega Nord esprimo solidarietà, purtroppo inutile, alla famiglia dell'ispettore Raciti**,** assassinato da un delinquente, frutto di una società senza valori e pervasa dal buonismo indiscriminato e permissivo. Ma tra pochi giorni ci saranno altri morti che cancelleranno il ricordo di oggi per essere a loro volta cancellati dalle trombe del calcio, amplificate dalla televisione, anche da quella di Stato. Solidarietà anche alle forze dell'ordine, per quanto serve. Lei sa, credo, Ministro, quanti agenti delle forze dell'ordine sono impegnati ogni settimana per tentare per tentare di garantire la sicurezza alle manifestazioni sportive e credo per il 99 per cento alle partite di calcio. Dati fornitici dalle dalle forze dell'ordine dicono che ammontano a circa 70.000 unità settimanali, per un costo di circa 5 milioni di euro a settimana. Moltiplichiamoli per le settimane del campionato di calcio e vedremo anche che cifra ne esce. Tutto questo a carico delle tasche dei cittadini italiani, perché le società di calcio, che a loro volta finanziano i gruppi di ultras, non spendono una lira per garantire, neppure all'interno delle loro strutture, un briciolo di sicurezza. E gli agenti delle nostre forze dell'ordine non hanno alcuna tutela perché, quando dovessero effettuare perquisizioni, sappiamo benissimo che ciò è possibile solo in presenza di un mandato. E quindi le denunzie fatte dai perquisiti spesso si ritorcono a titolo personale sugli agenti delle forze dell'ordine. Credo tutti conoscano - e qualcuno finge di non sapere il malessere e la frustrazione che li pervade; malessere e frustrazione dovuta al fatto che, dopo interminabili turni massacranti, non soltanto, per fortuna, per mantenere l'ordine a un gioco (quello che dovrebbe essere un gioco), rivedono dopo pochi giorni lo stesso delinquente che hanno catturato per strada, come se lo rivedono per strada tutti i nostri concittadini. Lo sport, però, signor Ministro, non è la causa di quanto sta succedendo in Italia, è uno dei tanti sintomi di questa società: il calcio ormai credo sia rimasto l'unico simbolo riconosciuto, molto più delle istituzioni, molto più del senso di appartenenza, molto più purtroppo anche della famiglia. Il problema è perché la nostra società sta diventando così. Forse lo possiamo capire, tra le altre cose, stando all'uscita delle scuole, dove spesso non si riconoscono gli insegnanti dagli allievi, né per come sono vestiti, né per come si comportano, né per l'anarchia che pervade tutto, partendo anche da quello che dovrebbe essere il primo inizio di conoscenza delle regole civili, quali le nostre scuole. Forze dell'ordine sottratte - 70.000 alla settimana, abbiamo detto - dalle strade. Questi agenti, poi, devono fare i recuperi; hanno delle turnazioni massacranti. E tutto questo si ripercuote sull'assenza nel nostro territorio delle forze dell'ordine per una media, calcolata da un rapporto del Ministero dell'interno, che dice che nel Lazio ci sono dieci rappresentanti delle forze dell'ordine ogni 1.000 cittadini; in Lombardia tre

quasi esattamente le stesse cose che ci sentiamo dire noi; ma l'aveva fatta la Lega, la Lega razzista, e la Lega non deve essere ascoltata, non può partecipare alla gestione della sicurezza del Paese. Occorre, credo, ripristinare anche la commissione degli affari interni, che in qualche modo cercava di coordinare i lavori. Ma mi chiedo, signor Ministro, come potete voi convivere con personaggi che affermano «ultras o poliziotto pari sono». E quando un giornalista oggi - sto parlando di agenzie - chiede a questo vostro collega: «Anche la maggioranza l'ha criticata?», «Certo, hanno paura. Il centro‑sinistra, invece di zittire quelli dell'opposizione, come qualcuno si è degnato di fare, li rincorre dicendo: «massima solidarietà alle forze dell'ordine». Si mettono a fare i più realisti del re». Sto parlando di un vostro collega che, se si mettesse le mani in tasca, ci troverebbe ancora i buchi nelle fodere, perché ci metteva bulloni e sampietrini, sto parlando del deputato Caruso. Non riesco a capire come possiate pretendere di essere credibili in quest'Aula semideserta, ma, soprattutto, se le nostre parole dovessero uscire nel mondo reale, dove vivono coloro che si illudono di essere rappresentati

che non stiamo lavorando, che stiamo soltanto aspettando che voi riusciate a coagulare in pochi giorni il numero di senatori necessario in quest'Aula per avere poi il voto di fiducia. Quale credibilità possiamo immaginare di avere partendo da questi presupposti? Vedete, signor Presidente, signor Ministro, il Governo, la Camera e il Senato dovrebbero dimostrare con i fatti di essere la voce del Paese. Con un guizzo di dignità, di cose concrete. Non mi sembra che siamo nelle condizioni di poterci riscattare con quanto succede per le strade. A noi dispiace un po' per gli italiani, signor Presidente, che hanno bocciato la legge sulla riforma federale dello Stato, ma vi assicuro che la Lega Nord brucerà le proprie energie solo per la sua terra, per il Nord. Senatore Pirovano, per quanto riguarda il lavoro, devo dirle che la mia preoccupazione è solo quella di organizzare, in rapporto con l'altra Camera, anche i lavori del Senato. Quindi, questa

Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, innanzi tutto è doveroso, ed è con profondo sentimento anche a nome dell'UDC, rivolgere un pensiero solidale e commosso a Filippo Raciti e alla sua famiglia, dalla quale abbiamo ricevuto tutti una testimonianza e, vorrei dire, una lezione esemplare. Va altresì manifestata profonda solidarietà alle forze di polizia, che vengono esposte ripetutamente e in più circostanze a rischi, e quando non a rischi ad inconvenienti e ad incomprensioni, che alimentano talvolta uno spirito di carattere negativo. Lei, signor Ministro, ha esposto, con la precisione e vorrei dire con l'acribia che la contraddistingue, innanzi tutto i fatti. Lo ha fatto anche riscattando l'esposizione rispetto al rischio del mattinale di polizia, con un certo *pathos*, che mi ha ricordato Gianni Brera. Mi consentirà subito, però, un'osservazione che non può non essere fatta: quella partita non andava giocata. Non basta dire che ci si è messo pure il diavolo con il ritardo con cui sono arrivati a Catania i quattro pullman. Quella partita, al di là di ciò che richiedeva la Lega calcio, non andava autorizzata. Noi abbiamo un ordinamento in questo Paese che mette in testa, al livello periferico e provinciale, al prefetto ‑ nel caso di Catania è un prefetto che merita ogni apprezzamento e stima ‑ le responsabilità dell'ordine pubblico: tutto faceva temere che accadesse qualcosa. Il tutto non si riporta soltanto ‑ vi farò qualche cenno ‑ alle spiegazioni della grande rivalità, che sta sullo sfondo anche di questa vicenda, tra Catania e Palermo, tra due squadre di calcio che dovrebbero festeggiare con la terza la prima volta in cui tre squadre di calcio siciliane si trovano tutte e tre in serie A. A. A Catania c'era quanto bastava per lasciare temere che potesse accadere un incidente indovinabile. Ma anche indominabile ‑ ecco la seconda osservazione se il dispiegamento delle forze di polizia negli stadi e attorno agli stadi continua ad avvenire (lo dico con profondo rispetto e riconoscenza) soltanto in termini di schieramento di forza, avendo rinunciato a svolgere quelle azioni aprioristiche di prevenzione che talvolta potrebbero essere molto più efficaci, avendo rinunciato a svolgere quell'opera di individuazione, di *intelligence*, si dice, che permette innanzi tutto di conoscere e di circoscrivere le persone dalle quali può venire l'insidia e il pericolo. Sappiamo tutti che nelle curve, dovunque (il problema non è solamente Catania), non si raccolgono soltanto persone perbene o giovani perbene: si raccolgono anche altri elementi ed altri soggetti; è temibile perciò che ci sia una compenetrazione che rappresenti un pericolo. Ho il dovere allora, per non rendere questo confronto con le dichiarazioni del Ministro soltanto di maniera, di fare le osservazioni che ho fatto.

in questi giorni, abbiamo dovuto ascoltare tanti interventi opportuni quanti inopportuni. Con il tentativo di spiegare gli eventi oltre lo spiegabile non si perviene al punto fondamentale al quale si deve arrivare; e il punto fondamentale al quale si deve tendere innanzi tutto esclude ogni forma di giustificazionismo. Questa forma di giustificazionismo è incombente pure quando ci si abbandona ad esercitazioni letterarie (ve n'è una su un quotidiano molto autorevole oggi che riporta addirittura la rivalità ai greci e ai fenici, agli albanesi e ai romani), di guisa che non si perviene al punto centrale al quale invece si deve mirare. Noi, la nostra società, la società italiana, non meno di altre società europee, siamo attraversati da una profonda crisi morale, che è determinata dalla mercificazione di tutto (anche io faccio letteratura); c'è stata in questi anni una mostruosa mercificazione del calcio, per cui il calcio da sport è diventato anche altro. Dobbiamo affrontare questo problema nei termini e nei modi in cui uno Stato si occupa anche delle questioni di moralità pubblica. Sarei, per esempio, molto convinto che, se il Ministro delle finanze si desse da fare attorno anche alle dichiarazioni dei redditi dei giocatori, non farebbe male, in maniera tale da introdurre elementi anche di demitizzazione di questo mondo.

Una delle prime reazioni del Ministro è stata quella di affermare: «Non manderò più le forze di polizia negli stadi». Capisco che questa possa essere una dichiarazione che nel momento...

Innanzitutto facciamolo rispettare compiutamente. Dal decreto Pisanu in poi si può vedere che cosa, in termini ulteriormente restrittivi, si debba fare, ma teniamoci sul terreno delle cose concrete. Il comportamento del Governo allora non deve essere elusivo di una precisa responsabilità, che è anche quella di lasciar riprendere il calcio senza interruzioni, che non avrebbero alcun significato e non porterebbero ad alcun risultato.

innanzitutto vorrei esprimere il cordoglio sincero del Gruppo di Rifondazione Comunista‑Sinistra Europea alla famiglia Raciti per la perdita che ha subìto e il nostro profondo dispiacere per una vita spezzata, per di più in un modo così futile e così gratuito. Ho ascoltato con attenzione e interesse la ricostruzione del Ministro dell'interno e l'ho anche in gran parte apprezzata, ma vorrei esprimere in questo intervento considerazioni di carattere più generale e anzitutto un certo profondo mio scetticismo. Sono decenni che si discute in questo Paese del problema della violenza negli stadi; sono anni che si susseguono incidenti, devastazioni, disordini, morti. Dal 1989 ad oggi sono state varate cinque leggi speciali. Mi permetto, da questo punto di vista, di dubitare della nostra capacità e possibilità d'intervento, al di là dei

una grande industria dello spettacolo, che produce non solo profitti, ma immaginari e che determina in questo modo un'influenza culturale profonda anche sui comportamenti di milioni di persone, è molto difficile pensare a come la politica possa intervenire per affrontare un tale problema. È più facile ‑ lo dico paradossalmente ‑ mettere in discussione in Italia il capitalismo che non il sistema del calcio. Questa è la prima constatazione amara che faccio in questa sede. Ne ho una prova lampante nelle recentissime esternazioni non di un ultrà, non di un passante qualunque, ma di uno dei massimi responsabili della nostra organizzazione calcistica, il presidente della Lega calcio, Antonio Matarrese, il quale ha dichiarato non non solo che lo spettacolo doveva continuare, ma che questi sono i prezzi che lo spettacolo del calcio non può non pagare. Ci sono dei prezzi da pagare, dei danni collaterali, dei morti che dobbiamo prevedere nei nostri bilanci. quasi lo stesso linguaggio che si adopera in guerra. Ed è questa, a mio parere, la grande difficoltà che gli eventi di Catania ci propongono. Bisogna capire come intervenire, perché certo qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna tentare, qualche intervento immediato va attuato. Io spero vivamente che il pacchetto di provvedimenti che il Governo ha varato e che presto sarà sottoposto al voto di quest'Aula non faccia la fine delle

il tifo, gli ultrà e le organizzazioni dei tifosi. Sappiamo piuttosto che dentro il mondo delle curve, dentro il mondo dei tifosi organizzati

diventa stabile, identitario, concorre alla diffusione di disvalori profondi e fa della violenza e anche, certo, della lotta alle forze dell'ordine un elemento di identità

avviare una riflessione di fondo oltre l'emergenza, oltre gli eventi da cui siamo scioccati, oltre il momento specifico? Credo che ciò sarebbe molto utile a tutti.

signor Ministro, e non credo nemmeno serva un vero e proprio ossimoro quale la flagranza differita, che non a caso l'intera Unione dei penalisti giudica inammissibile sul terreno strettamente giuridico. Servono certamente pene

organizzato il suo possibile significato di momento di aggregazione su valori che non siano la distruzione dell'altro, la sopraffazione e la violenza, addirittura come atti di celebrazione della propria identità.

Tale apprezzamento si tradurrà nella leale disponibilità a collaborare nei lavori per la conversione del decreto-legge che vi apprestate a varare, nella misura in cui gli articoli del gli articoli del decreto saranno coerenti con questi propositi, riservandoci, ovviamente, l'esame analitico delle singole norme, magari al netto di annunci inutili - non so bene, infatti, cosa sia l'Osservatorio sui giornalisti sportivi - e anche di sovrabbondanze sociologiche. I decreti attuativi della legge Pisanu vanno applicati per intero da tutti, nel più breve tempo possibile, perché sono norme dello Stato e perché la loro configurazione è frutto di un percorso a suo tempo condiviso con ANCI, CONI, Federazione giuoco Calcio e con tutte le Leghe Oggi nessuno di questi soggetti e nessuno dei Comuni e delle società che da questi soggetti sono rappresentati, può dire di non essere stato consultato; nessuno può dire di aver ricevuto imposizioni dall'alto e ciò vale non solo per le società, delle quali non condivido la generalizzata criminalizzazione, ma vale anche, nella stessa misura, per i Comuni proprietari di quasi tutti gli impianti sportivi.

fosse chiamato a votare un ordine del giorno simile a quello per la base USA di Vicenza nel quale si dicesse: «Ascoltate le dichiarazioni del Governo e in particolare del ministro Amato, le approva»,

perché con la medesima chiarezza dell'onorevole Caruso dico che non è vero che l'omicidio di un poliziotto è equiparabile alla morte di un ultrà o di un esponente dell'antagonismo: non è vero! Su questo non ci possono essere né incertezze, né sfumature: Carlo Giuliani a Genova è morto perché voleva colpire un carabiniere con un estintore, l'ispettore Raciti a Catania è morto perché voleva difendere la sicurezza di tutti noi, e se qualcuno si ostina a non capirlo, al punto da dedicare una sala in questo Senato a Carlo Giuliani, le persone di buon senso percepiscono l'aggressione ad un poliziotto come l'aggressione a se stessi e alla comunità che quel poliziotto tutela. Gli eroi non sono quelli con l'estintore in mano: gli eroi sono quelli che, nonostante lo stipendio basso, i giudici che scarcerano, le società e i comuni inadempienti, indossano la divisa ed escono di casa, come lei stesso ha ricordato, Ministro, senza essere certi di tornarci. Ma Francesco Caruso non è estemporaneo, perché in fondo ha ribadito ciò che è contenuto nel programma dell'Unione, che anche voi, signor Ministro e signor Presidente, avete sottoscritto,

anche «regole per migliorare la riconoscibilità degli operatori delle forze dell'ordine nel corso delle operazioni di ordine pubblico», che è come dire «chi dei poliziotti riesce a sfuggire all'aggressione durante gli scontri sappia che lo andiamo a trovare sotto casa». Allora la nostra disponibilità c'è, ma sarà tanto maggiore quanto più reale sarà la vostra presa di distanza da questo programma infantile ed estremista; e se l'estremismo era la malattia infantile di una cosa che la storia grazie a Dio sta cancellando, la violenza negli stadi è il segno dell'infantilismo di frange sociali troppo viziate e troppo stupide, frange sociali i cui vizi e la cui stupidità possono essere contrastate solo con l'applicazione rigorosa di una legge finalmente seria. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, lei a mio avviso ha fatto bene ad introdurre la sua informativa con una breve ma significativa riflessione sulle diverse forme di violenza che si addensano o condensano ed esplodono negli stadi. Noi dobbiamo prendere atto che il sistema calcio è diventato di per sé un incubatore di violenza e che alcune delle sue componenti non si oppongono alla violenza e talvolta persino la assecondano. E dunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, è di questa violenza non ostacolata o addirittura facilitata che dobbiamo occuparci. Condivido l'impostazione generale che il ministro Amato ha dato al problema e naturalmente attendo di vedere i provvedimenti che il Governo si accinge a prendere prima di formulare giudizi puntuali. Dico subito, però, che condivido totalmente il proposito di garantire immediatamente la piena applicazione dellenorme esistenti. Mi permetto di ricordare che, in sede di prima applicazione, e di applicazione parzialissima, nel campionato 2005-2006, quelle norme hanno consentito di ridurre della metà la violenza complessiva negli stadi, nonostante soltanto cinque o sei stadi su 31 avessero applicato quelle norme, specialmente per quanto riguarda l'apprestamento delle infrastrutture di sicurezza al di fuori e all'interno degli stadi medesimi.

Spendono cifre enormi, inaudite, per gli ingaggi ai campioni, ma non sono disposte o non si sono dimostrate finora disposte a spendere cifre relativamente modeste per garantire la sicurezza degli spettatori, delle forze di polizia e degli stessi calciatori*. Sono dunque necessarie norme che costringano le società sportive a investire. Esse hanno avuto un anno e mezzo di tempo per realizzare queste infrastrutture e non lo hanno fatto. Ieri sera, in una trasmissione televisiva, il presidente del Catania ha detto che in tre mesi è in grado di fare ciò che non è stato fatto in un anno Sono d'accordo con lei, signor Ministro, sul divieto della vendita in blocco dei biglietti destinati agli ospiti, perché le trasferte costituiscono l'occasione per una moltitudine di reati e violenze. Attenzione: a Catania gli ospiti erano 500 ed erano arrivati ordinatamente all'inizio del secondo tempo. Nonostante ciò, le violenze a Catania ci sono state e sappiamo in

intrecci perversi tra società sportive, tifoserie e anche alcuni ambienti politici, cosicché possiamo dire che spesso la violenza nelle curve è, più o meno consapevolmente, sovvenzionata dalle associazioni sportive e da coloro che si dichiarano sportivi «ultras». Inoltre, sono d'accordo sull'ampliamento dell'arresto in flagranza differita a quarantotto ore ‑ come io stesso avevo proposto ‑ e credo che la norma vada stabilizzata. Capisco le obiezioni che vengono mosse ‑ e sono sincere ‑ da giuristi illustri in questa e nell'altra Aula del Parlamento. Si deve però considerare che quella norma ha avuto uno straordinario effetto didissuasione sui violenti e che abbandonarla oggi significherebbe letteralmente abbassare la guardia.

e lo sono ‑ i principali bersagli della violenza negli stadi è a loro che dobbiamo rivolgere le maggiori attenzioni.

Quindi, se non ci pensano costoro, ci pensi lo Stato, ci pensi il Parlamento, garantendo innanzitutto alle forze dell'ordine migliori condizioni di lavoro e di vita, ma introducendo anche norme che, tutelando il loro lavoro, tutelino la sicurezza di tutti. Che cosa osta, ad esempio, all'introduzione di un'aggravante specifica per resistenza a pubblico ufficiale, almeno quando questa resistenza si realizzi in contesti di particolare rischio? Che cosa ci impedisce di approfondire la possibilità di intravedere un reato associativo per gruppi di sportivi che, in partenza, si organizzino per compiere molteplici atti di violenza? Una riflessione parallela è stata fatta in passato per gli anarco‑insurrezionalisti, e magistrati illuminati hanno risolto positivamente la situazione individuando il reato associativo, anche laddove gli associati, per loro stessa scelta ideologica e programmatica, si dichiaravano individualisti. Dobbiamo costringere, con misure dirette e indirette, le società sportive a spendere di più per la sicurezza. Ma che cosa ci vuole a capire che la testa di un poliziotto o di un carabiniere vale quanto la testa di un capocannoniere? Che cosa ci vuole ad assumere una valenza morale minima per la tutela dell'ordine e della sicurezza nei nostri stadi? Ho apprezzato molto, signor Ministro, la fermezza con cui lei ha difeso le forze dell'ordine; altro che dottrina Caruso. Ci vuole ben altro che le compiacenze ideologiche e politiche che hanno portato l'onorevole Caruso a sedere in Parlamento. Naturalmente noi condividiamo il proposito del Governo di guardare alla privatizzazione degli stadi e alla possibilità di coinvolgere pienamente le società sportive per garantirne la sicurezza. Ma il punto su cui dobbiamo concentrare oggi tutti gli sforzi è la sicurezza negli stadi, la creazione delle condizioni appropriate perché le forze dell'ordine possano svolgere il loro lavoro con la massima efficacia e il minore rischio possibile, altrimenti le cerimonie e le lacrime di questi giorni, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tramuteranno in un'indegna e disumana commedia. Signor Ministro, il mio Gruppo la ringrazia per la sua presenza in Senato e la sua informativa,

ricordare, seppure molto brevemente, che il cammino della democratizzazione delle forze di polizia in questo Paese ha condotto, nel corso dei decenni,

dobbiamo continuare ad attingere nel momento in cui episodi come quelli di cui stiamo discutendo segnalano una vera e seria difficoltà, seria difficoltà, per la quale noi abbiamo il dovere innanzitutto di ringraziare gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Tale difficoltà deve portarci però anche a riflettere su altro, su una certa idea primitiva della regolazione di legalità che pure, negli interventi di oggi,

Invece non si può, in una società complessa, in una democrazia complessa e in un mercato complesso che lega insieme il valore dello sport agli interessi commerciali così forti e dominanti delle società calcistiche e dell'intero mercato che al calcio si collegano, dimenticare che il compito della regolazione della legalità non può essere caricato esclusivamente sulle spalle dei poliziotti e delle poliziotte italiane e dei carabinieri e delle carabiniere italiane. Lo dico legislatura ho condiviso con l'ex ministro Pisanu la fatica della costruzione del provvedimento da cui oggi partiamo e continuiamo ad attingere la forza per raggiungere misure che coerentemente si muovano e per le quali ringrazio il ministro Amato

stata la sconfitta in Aula perché la forza delle società calcistiche è stata tale da impedire che su di esse gravasse almeno in parte il costo della sicurezza negli stadi.

sottolineo che i ragazzi con il passamontagna organizzati che hanno devastato, picchiato, distrutto ed ucciso sono figli di quella città. Non lo affermo con commozione di madre, ma con la durezza di chi è chiamato a compiti di responsabilità pubblica. Se sono figli nostri e di quella città, non possiamo fare finta che non esistano e che siano figli di quella città e del suo disagio, delle sue difficoltà, delle sue periferie e della sua incultura. Ciò non vuol dire che la città sia solo loro, perché Catania - lo ripeto - è Filippo Raciti, è sua moglie, è tutti i cittadini catanesi che oggi hanno sofferto. Per fare questo, dobbiamo contrastare una

si mischi con il sacro e occupi il luogo del sacro, che vi sia mercato anche lì dove ci deve essere solo preghiera e raccoglimento. e raccoglimento. Al senatore Mantovano, che conosco da tanti anni, sottolineo che le morti sono tutte uguali; possono essere diverse le ragioni per le quali si muore, ma il valore della vita è identico.

Altrettanto non mi convincono completamente le dichiarazioni del signor Ministro. Per ragioni di tempo, mi limito a svolgere una sola considerazione. In ogni Paese civile, in ogni Paese europeo, vengono risarcite le famiglie dei tutori dell'ordine in tempi ragionevolissimi. Chiedo al signor Ministro di assumere un preciso impegno: che alle parole di solidarietà seguano i fatti di solidarietà. Quindi, fra tre mesi, chiederò al signor Ministro Ministro se è stato accreditato l'indennizzo alla famiglia Raciti e, nel frattempo, se è vero ciò che alcuni giornali hanno riportato, vale a dire che alla vedova Raciti perverrà una pensione di reversibilità di poco meno di 500 euro. Credo che il signor Ministro dell'interno, se ha veramente a cuore le forze dell'ordine, i tutori dell'ordine, soprattutto quelli che hanno dato la vita allo Stato, si ponga il problema di discutere di assegni di reversibilità non nel prossimo Consiglio dei ministri per le coppie di fatto, bensì per le vedove dei tutori dell'ordine.